ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. **Sull'ordine dei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 finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2024

Superato lo scoglio della revisione del quadro finanziario pluriennale, che è stata oggetto dell'ultimo Consiglio straordinario, una parte molto significativa delle discussioni in agenda di questa riunione verterà sui grandi temi di politica internazionale. Si partirà, naturalmente, dalla situazione in Ucraina, dalla risposta europea all'aggressione russa; insieme agli altri *leader* europei, ribadiremo ancora una volta il nostro sostegno all'Ucraina, un sostegno che ho voluto riaffermare a nome dell'Italia convocando la prima riunione dei *leader* del G7 sotto Presidenza italiana proprio da Kiev nel secondo tragico anniversario della brutale invasione russa e dell'eroica resistenza ucraina. Voglio cogliere l'occasione per rivendicare con orgoglio il ruolo che il nostro Governo ha svolto dapprima nel Consiglio del dicembre scorso per contribuire a sbloccare il negoziato per l'avvio del percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione europea e poi nel Consiglio straordinario di febbraio, per favorire una soluzione positiva proprio sulla revisione del quadro pluriennale finanziario, comprensivo di un adeguato stanziamento per l'Ucraina, ma anche di risorse fondamentali per affrontare alcune delle principali questioni di nostro interesse, dal sostegno alla competitività fino alla lotta all'immigrazione illegale. Non era una trattativa facile e probabilmente non avrebbe avuto questo epilogo se avessimo seguito i consigli di quanti, anche in quest'Aula, da tempo sostengono che non si debba dialogare con tutti, ma solamente con alcuni, in questa bizzarra idea di un'Unione europea distinta tra Nazioni di serie A e Nazioni di serie B. Pare che la linea vincente e più utile all'Italia, oltre che alla comune causa europea e occidentale, sia invece quella sostenuta da chi, come la sottoscritta, ha sempre considerato tutti i *partner* europei degni di rispetto e di considerazione. *(Applausi)*. Sempre in tema di Ucraina, in questi giorni si è molto discusso della proposta avanzata in particolare dalla Francia circa un possibile intervento diretto di truppe di Nazioni dell'Unione europea in Ucraina. Approfitto per ribadire anche in quest'Aula, come fatto ampiamente anche dal ministro degli affari esteri Tajani, che la nostra posizione non è favorevole in alcun modo a questa ipotesi, che consideriamo foriera di un'*escalation* pericolosa da evitare invece ad ogni costo. *(Applausi)*. Spero che questo Parlamento sia compatto nel rispondere con noi sul punto. Come ho più volte ribadito anche in quest'Aula, sostenere l'Ucraina vuol dire tutelare il nostro interesse nazionale e il nostro impegno rimane finalizzato su tutto alla creazione delle condizioni per una pace giusta, duratura, rispettosa della dignità della Nazione aggredita. Ogni nostra azione ha prevalentemente questo scopo e mi stupisce - ma forse non dovrebbe - che proprio chi più si riempie la bocca con la parola «pace» abbia contestato la sottoscrizione da parte italiana di un accordo pluriennale di cooperazione e di sicurezza con l'Ucraina. La cooperazione di lungo termine sulla sicurezza che abbiamo offerto, infatti, riguarda più la pace che non il conflitto. La ragione è semplice: gli ucraini fanno presente che un ostacolo fondamentale a qualsiasi possibile negoziato sta nel fatto che fin qui la Russia ha sistematicamente violato gli accordi sottoscritti e il diritto internazionale. Basti pensare che dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, con il *memorandum* di Budapest del 1994, Kiev ha consegnato a Mosca le numerose testate atomiche in suo possesso in cambio del rispetto dell'inviolabilità dei confini ucraini. A nessuno sfugge che una potenza atomica non sarebbe stata invasa dai russi nel 2014 e poi di nuovo nel 2022, come invece è accaduto in violazione di quel *memorandum*. Pertanto, come ci si può ragionevolmente sedere a un tavolo di trattative con qualcuno che non ha mai rispettato gli impegni assunti? Eco perché gli impegni internazionali di sicurezza in favore dell'Ucraina sono il prerequisito indispensabile a qualsiasi accordo di pace tra Ucraina e Russia. Non si tratta, come qualcuno prova oggi a raccontare, dell'impegno a fornire armi per i prossimi dieci anni; si tratta, invece, di un'intesa multidimensionale che fa seguito ad analoghi accordi sottoscritti da altri Stati europei e occidentali, che riguarda una cooperazione a 360 gradi, compresa la ricostruzione, l'assistenza umanitaria, una rafforzata collaborazione politica e di sicurezza, come è naturale che avvenga nei confronti di uno Stato che ha avviato il percorso di adesione all'Unione europea. Detto questo, l'Italia saluta con favore l'ingresso definitivo della Svezia e della Finlandia nell'Alleanza atlantica e condanna ogni atteggiamento aggressivo da parte della Federazione Russa nei confronti di questi due Paesi amichi e alleati, così come nei confronti dei Paesi baltici. Allo stesso modo, ribadiamo la nostra condanna allo svolgimento di elezioni farsa in territorio ucraino e alle vicende che hanno portato al decesso in carcere di Aleksei Navalny, il cui sacrificio in nome della libertà non sarà dimenticato.

Il Consiglio europeo tratterà naturalmente anche dell'altro drammatico conflitto in corso, quello tra Israele e Hamas. Come sapete, sono reduce da una missione in Egitto (sulla quale tornerò anche più tardi), nel corso della quale, insieme alla Presidente della Commissione europea e a diversi *leader* europei, abbiamo incontrato il presidente al-Sisi, con il quale abbiamo discusso della situazione a Gaza e della necessità di continuare a lavorare senza sosta per evitare un'estensione del conflitto che, come ho già detto anche in quest'Aula, avrebbe conseguenze potenzialmente inimmaginabili. Siamo fortemente impegnati affinché il Consiglio europeo possa adottare una posizione autorevole sulla crisi e sul contributo che l'Europa può offrire alla soluzione. Ribadiremo ancora una volta la nostra ferma condanna della brutale aggressione perpetrata da Hamas il 7 ottobre scorso e ribadiremo la richiesta di un immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, perché non possiamo dimenticare chi non possiamo dimenticare chi è stato a scatenare questo conflitto, massacrando civili inermi, donne e bambini compresi, e mostrando al mondo i loro corpi oltraggiati. È stato Hamas e lo sottolineo perché la reticenza che sempre più spesso si incontra nel ribadirlo tradisce un antisemitismo latente, ma dilagante, che ci deve preoccupare tutti. Ribadiremo anche che il legittimo diritto all'autodifesa di Israele deve esercitarsi con proporzionalità e nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Non possiamo restare insensibili di fronte all'enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte: prima del cinismo di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane. Ribadiremo la nostra contrarietà a un'azione militare di terra da parte di Israele a Rafah, che potrebbe avere conseguenze ancora più catastrofiche sui civili ammassati in quell'area. Riaffermeremo la necessità di assicurare la consegna in sicurezza degli aiuti umanitari e il sostegno all'iniziativa Amaltea per un canale marittimo da Cipro a Gaza, finalizzato alla consegna degli aiuti stessi, fermo restando naturalmente la necessità di aprire nuove vie terrestri che rimangono prioritarie. Confermeremo il nostro sostegno agli sforzi di mediazione portati avanti in particolare da Stati Uniti, Egitto e Qatar per un prolungato cessate il fuoco che possa consentire il rilascio incondizionato degli ostaggi e massicci aiuti umanitari alla popolazione civile. Proprio sul piano umanitario prosegue l'incessante lavoro dell'Italia a favore della popolazione civile di Gaza, che, dopo l'invio della nave ospedale Vulcano e le iniziative congiunte con i Paesi del Golfo in particolare, vede ora anche l'arrivo di bambini palestinesi nei nostri principali ospedali pediatrici - che voglio ringraziare - per poter essere curati. Il Governo italiano, in ultimo, saluta con favore il cambio di *leadership* in seno all'Autorità nazionale palestinese, che ci auguriamo possa consentire di rilanciare la soluzione a due Stati, sulla quale continuiamo a ritenere prioritario avviare iniziative concrete e l'Europa in questo può e deve, dal nostro punto di vista, giocare un ruolo da protagonista. Come sappiamo, le conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas si ripercuotono in modo diretto su tutto il Medio Oriente e la nostra preoccupazione va anche a quanto sta avvenendo nel Mar Rosso. Permettetemi in primo luogo di rivolgere un pensiero di sincera gratitudine alla Marina militare italiana *(Applausi)* e all'equipaggio della nave Duilio, e all'equipaggio della nave Duilio, che si trova in questi giorni nelle acque prospicienti il Mar Rosso, impegnata in una missione dall'alto potenziale di rischio per assicurare la sicurezza e la libertà di navigazione alle nostre navi commerciali. In questi giorni la nave Duilio ha dovuto neutralizzare più di un attacco portatole da droni Houthi, lo ha fatto con prontezza ed efficacia, così come, sempre con prontezza ed efficacia, operano le nostre Forze armate. È anche per questo che proprio all'Italia è stato assegnato il comando tattico dell'operazione europea Aspides, deliberata con tempestività dalle istituzioni europee soltanto poche settimane fa. Tutti noi sappiamo quanto le minacce e le operazioni degli Houthi facciano parte di un disegno più vasto, che vede purtroppo l'Iran impegnato in prima linea nel sostenere non soltanto gli Houthi, ma anche Hamas e Hezbollah, nonché a fornire di droni le operazioni russe in Ucraina. Sappiamo anche quanto sia importante quel tratto di mare per i nostri interessi economici e geostrategici e quanto sia concreto il rischio che i maggiori costi sostenuti dalle nostre compagnie di navigazione finiscano non soltanto per comprometterne la competitività, ma anche per scaricarsi sul prezzo finale delle merci, portando a un nuovo aumento dei costi per i consumatori proprio ora che l'inflazione sta finalmente scendendo e l'Italia si distingue per l'inflazione più bassa registrata tra le economie del G7. La vicenda del Mar Rosso ci dimostra anche quanto siano importanti una chiara visione europea a tutela dei nostri interessi e una politica di sicurezza e difesa all'altezza delle nostre ambizioni e delle nostre esigenze difensive. Nel prossimo Consiglio ci sarà infatti un dibattito, quanto mai urgente e delicato, sulla sicurezza e sulla difesa europea. Voglio dire con chiarezza che l'Italia è pronta a fare la propria parte nello sviluppo della strategia europea per l'industria della difesa, presentata alcuni giorni fa dalla Commissione. E qui francamente, penso, signori, che occorra smettere di essere ipocriti sul tema, perché le accuse di un'eccessiva ingerenza americana e gli strali contro una seria politica di difesa nazionale ed europea camminano curiosamente sempre insieme, ma insieme non stanno. Se chiedi a qualcuno di occuparsi della tua sicurezza, devi prendere in considerazione l'ipotesi che quel qualcuno avrà grande voce in capitolo quando si tratterà di discutere di dinamiche internazionali. Dunque, spendere in difesa significa investire nella propria autonomia, nella propria capacità di contare e decidere, nella propria possibilità di difendere al meglio i nostri interessi nazionali ed è la strada che segue qualsiasi Nazione seria, ma è la strada che deve seguire anche l'Europa, se vuole essere seria. Per questo sarà necessario approfondire il tema delle risorse che servono, anche a livello europeo, per fare un salto di qualità nel settore della difesa e l'Italia vuole essere tra i protagonisti di questo dibattito e tra quanti promuovono anche soluzioni innovative per dotarci di finanziamenti necessari. Rivendichiamo da sempre la necessità che la NATO sia composta da due colonne, una americana e una europea, con pari dignità e pari peso, ma questo significa anche rispettare i vincoli previsti e sottoscritti, dotarsi di adeguata forza industriale e capacità di deterrenza, senza la quale non potrà esserci né sicurezza né libertà per i nostri popoli. Sì, la libertà ha un costo, la sovranità ha un costo e non credete a chi vi dice che tutto può esservi concesso gratuitamente. *(Applausi)*. Il risultato spesso, come si è visto, è che si paga molto di più. Le esigenze di sicurezza e difesa dell'Unione europea sono strettamente connesse anche al tema dell'allargamento dell'Unione, o meglio della riunificazione dell'Europa, come preferiamo definirla. Come sapete, l'Italia ha investito molto su questo processo, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Sosteniamo il percorso di avvicinamento all'Unione europea per tutti i candidati, sia quelli orientali sia quelli dei Balcani occidentali. In questo quadro siamo pronti a sostenere ancora una volta, alla luce della raccomandazione contenuta nel relativo rapporto della Commissione, l'apertura dei negoziati di adesione per la Bosnia Erzegovina. Si tratta di una decisione che siamo convinti possa portare a ulteriori e decisivi progressi da parte di Sarajevo nel percorso di riforme verso l'Unione europea. Del resto, abbiamo già visto come la concessione a dicembre del 2022 dello *status* di Paese candidato alla Bosnia Erzegovina l'abbia portata a realizzare in poco più di un anno un numero di riforme superiore a quanto fatto nei precedenti dieci anni. Il Consiglio prossimo sarà anche l'occasione per fare il punto sulla risposta europea in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di esseri umani, un *dossier* che ormai viene calendarizzato a ogni riunione su esplicita richiesta italiana, per tenere monitorati i progressi grazie a comunicazioni puntuali da parte della Commissione. Come sapete, sono reduce da una missione molto significativa in Egitto, insieme alla presidente della Commissione europea von der Leyen, al presidente di turno del Consiglio europeo De Croo, al presidente cipriota Christodoulidis, al cancelliere austriaco Nehammer, al primo ministro greco Mitsotakis. Si è trattato di un vertice molto produttivo che si è concluso con la firma di una dichiarazione congiunta UE-Egitto, propedeutica a un accordo di partenariato strategico e globale che segna indubbiamente un salto di qualità nelle relazioni con un *partner* fondamentale del Mediterraneo. Approvvigionamento energetico, sicurezza, capacità di mediazione nel conflitto mediorientale, gestione dei flussi migratori sono i principali punti di un documento comune che fornisce un nuovo quadro di riferimento nei rapporti con questo importante vicino. Sapete che l'Italia si è molto impegnata per esportare il modello Tunisia anche ad altre Nazioni africane del Mediterraneo e sapete anche che l'Italia si era già mossa in questa direzione a livello bilaterale, rilanciando la cooperazione con l'Egitto nell'ambito del Piano Mattei; cooperazione che domenica scorsa abbiamo ulteriormente concretizzato con la firma di diverse intese bilaterali. Grazie a questa rinnovata cooperazione e ai buoni rapporti coltivati abbiamo raggiunto l'importante risultato della scarcerazione di Patrick Zaki, ma, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la ricerca della verità sul caso di Giulio Regeni *(Applausi)*, come dimostra il processo in corso in Italia, che il Governo segue con molta attenzione e rispetto al quale ci siamo costituiti parte civile. Continuiamo a ritenere che la strada di una cooperazione di lungo periodo strutturata con le Nazioni africane e mediterranee sia anche lo strumento più efficace per costruire una soluzione strutturale al problema migratorio e l'accordo UE-Tunisia, fortemente promosso dal Governo italiano, che oggi sta dando i suoi frutti proprio sul fronte migratorio, dimostra come la strada intrapresa sia quella giusta. Gli ultimi dati forniti da Frontex certificano infatti un calo di arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale di circa il 60 per cento nei primi mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una sensibile diminuzione proprio di quelli provenienti dalla Tunisia. Aggiungo l'importante dato che riguarda la drastica riduzione della rotta proveniente dalla Turchia, che negli anni scorsi ha rappresentato una delle maggiori criticità per l'Italia. Siamo quindi particolarmente orgogliosi che il modello di cooperazione rafforzata con i Paesi del Mediterraneo allargato, su cui il nostro Governo ha investito tante energie, in questi mesi diventi il paradigma di riferimento anche per l'Unione europea nel suo complesso. E mi auguro che non ci siano opposizioni ideologiche o strumentali lungo il percorso che ci porterà all'attuazione dell'accordo con l'Egitto, come purtroppo abbiamo ancora una volta dovuto constatare alcuni giorni fa proprio sulla Tunisia. Sul fronte migratorio, però, non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia. L'arrivo della bella stagione può incoraggiare i trafficanti di esseri umani nel provare a intensificare i loro traffici. Per questa ragione, è fondamentale attuare pienamente il piano d'azione in dieci punti presentato dalla Commissione europea e attualmente in fase d'implementazione, così com'è importante allargare la cooperazione con i Paesi africani in tema di lotta alle reti di trafficanti anche oltre i confini europei. È la ragione per la quale Africa e migrazioni saranno anche al centro della Presidenza italiana del G7 e il nostro duplice obiettivo è, da una parte, quello di aumentare gli sforzi sul Continente africano e, dall'altra, quello di lanciare un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. Il nuovo approccio a carattere onnicomprensivo e multidimensionale alla sfida migratoria, adottato su spinta italiana dall'Unione europea, è stato ben descritto nella comunicazione pubblicata dalla Commissione in vista del Consiglio, che tratteggia sviluppi e prospettive dell'azione continentale. Questo nuovo approccio viene confermato anche *pro futuro* in chiave di attuazione e rafforzamento di tutte le misure concordate, con una specifica forte attenzione alla prospettiva degli Stati membri mediterranei. un approccio ritagliato in tutte le sue componenti, anche e soprattutto sulle loro esigenze, cioè sulle nostre esigenze. Al Consiglio europeo promuoveremo un'ulteriore sottolineatura del carattere prioritario della dimensione esterna per una soluzione strutturale alla sfida migratoria, che rimane l'aspetto per noi assolutamente cruciale. Questo Consiglio europeo si occuperà - finalmente, lasciatemelo dire - anche di agricoltura. È stata una richiesta avanzata particolarmente dall'Italia, che siamo lieti sia stata recepita.

di intervenire a sostegno di un settore che è stato troppo a lungo dimenticato e oggetto di attenzioni non sempre benevole. La doppia crisi pandemia-guerra ha colpito anche le catene d'approvvigionamento alimentare e gravato le imprese agricole di un aumento dei costi fissi che ne ha ulteriormente ridotto la redditività. A questo si sono aggiunti, da un lato, l'appesantimento burocratico introdotto dalle misure d'inverdimento della politica agricola comune (PAC) e, dall'altro, l'accanimento ideologico di molte norme del *green new deal*, del pacchetto "Fit for 55" e della strategia "Farm to Fork". L'Europa si è così risvegliata con i trattori nelle strade, in prima battuta nei Paesi che avevano adottato ulteriori misure nazionali particolarmente penalizzanti per il settore, a cominciare dall'interruzione dei sussidi per il gasolio agricolo, scelta che invece non ha fatto l'Italia, che li ha prorogati. *(Applausi)*.

queste, a differenza delle loro colleghe omologhe di Francia, Germania, Belgio, Spagna, Olanda e di molti altri Paesi, non hanno partecipato alle manifestazioni. Rivendico con orgoglio che il nostro è stato sinora il Governo che più ha investito in agricoltura nella storia repubblicana *(Applausi)*, arrivando a stanziare, grazie alla tanto vituperata rimodulazione del PNRR, fino a otto miliardi per il comparto agricolo. Si tratta di una scelta strategica, alla quale si sono aggiunti in questi diciassette mesi di Governo molti altri importanti provvedimenti, dei quali questo Parlamento ha già avuto modo di discutere qualche settimana fa. L'ultimo intervento riguarda la questione dell'Irpef agricola, inserita, seppur marginalmente, anche in alcune piattaforme dei manifestanti: rivendichiamo la scelta di non esentare dal pagamento le imprese di maggiori dimensioni, che possono permettersi di pagarla, e quella di concentrare invece le risorse destinate al comparto agricolo a favore di chi ne ha davvero bisogno, non solo esentandolo dal pagamento dell'Irpef, ma anche con ulteriori misure di sostegno Soprattutto però gli agricoltori - e, con loro, i pescatori - sanno che fin dal primo giorno il nostro Governo in sede europea ha contrastato quella visione ideologica della transizione *green* che ha individuato proprio nell'agricoltore, nel pescatore e negli operatori economici che lavorano a contatto con la natura dei nemici da colpire in nome della guerra santa contro il cambiamento climatico. Per noi, invece, l'agricoltore è il primo ambientalista, è il bioregolatore per eccellenza, è il garante della nostra sicurezza alimentare, è colui che ha il maggiore interesse a preservare la natura, atteso che proprio dalla natura trae il suo reddito. Come tale, deve essere pienamente coinvolto nelle politiche di riduzione delle emissioni. *(Applausi)*. Se, infatti, lo graviamo di oneri insostenibili sul piano economico e burocratico, fino a far finire la sua azienda fuori mercato e a farlo chiudere, il giorno dopo quel pezzo del nostro ambiente rurale sarà abbandonato all'incuria e alla fine produrrà maggiori danni. *(Applausi)*. Su questo argomento, proprio il nostro Governo ha presentato un documento che è stato sostenuto da tutti i Ministri agricoli. Ora ci auguriamo che dalla discussione dei prossimi giorni possano scaturire indicazioni forti alla Commissione e al successivo consiglio Agrifish del 26 marzo, soprattutto in alcune direzioni. Abbiamo accolto con favore l'annuncio della Commissione di un ritiro definitivo della proposta legislativa in materia di agrofarmaci, che il Parlamento europeo prima ed il Consiglio poi, avevano bocciato. Ora è urgente, in primo luogo, intervenire sull'attuazione della Politica agricola comune. Penso che possiate convenire con me sul fatto che, quando tutti noi abbiamo sostenuto la vecchia PAC, il contesto era molto diverso da quello attuale. Non si era ancora verificato lo *shock* dell'invasione russa in Ucraina, in primo luogo. In secondo luogo, la Politica agricola comune che è stata votata era comunque una mediazione rispetto alle folli pretese dell'allora vice presidente Timmermans, che voleva una PAC ancora più sbilanciata verso le misure di inverdimento, tanto da voler ricomprendere al suo interno gli obiettivi di riduzione delle emissioni del *green deal*. Queste pretese non si materializzarono allora, ma si sono verificate successivamente, con la definizione degli ecoschemi e delle condizionalità verdi. Ed è proprio da quelli che si deve partire, semplificando al massimo le procedure, eliminando con effetto retroattivo l'obbligo di messa a riposo del 4 per cento dei terreni e l'obbligo di rotazione delle colture, che limiterebbe in maniera sensibile la produttività delle nostre imprese. La recente proposta della Commissione di ampia revisione della PAC va nella giusta direzione, riprendendo molte delle proposte italiane. Ora è importante lavorare rapidamente alla riforma, a partire dal prossimo Consiglio agricoltura e pesca di fine marzo. lavoriamo perché possano trovare spazio anche altre proposte italiane, come l'estensione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prevedendo comunque un incremento del regime *de minimis*, nonché una moratoria dei debiti delle imprese agricole. In questo contesto così difficile, è indispensabile rafforzare anche la nostra risposta alla concorrenza sleale dei Paesi terzi, affermando il principio di reciprocità; condurre i futuri negoziati sugli accordi di libero scambio, a partire da quello sul Mercosur, con una accresciuta attenzione al mondo agricolo; intervenire anche sulle importazioni agricole dall'Ucraina, affinché i sacrosanti sforzi che hanno portato a ripristinare i corridoi della *green initiative* siano orientati verso i Paesi terzi più bisognosi di grano e di altre materie prime e non producano ulteriore concorrenza al ribasso, a scapito dei produttori europei. Infine, dato anche questo molto importante, siamo ancora in una fase di asimmetria nella distribuzione del valore lungo le filiere, soprattutto in alcuni settori. Oltre all'opera di *moral suasion* che il Governo potrà svolgere tra tutti gli interlocutori, sarà importante rafforzare la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che potrà aiutare a garantire il giusto prezzo alle nostre imprese agricole. Infine, voglio cogliere l'occasione di questo dibattito parlamentare per condividere con voi la soddisfazione in merito all'esito del negoziato sul nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Sono fiera del risultato raggiunto e sono fiera del grande lavoro di squadra che è stato fatto dall'intero sistema Italia. Governo, imprese, associazioni di categoria, Parlamento nazionale, parlamentari europei di diversi schieramenti, col supporto dei nostri funzionari a Bruxelles, hanno remato tutti nella stessa direzione, per preservare un modello di eccellenza nell'economia circolare, che è stato costruito nel corso degli anni con il contributo straordinario di tante nostre imprese e dei cittadini italiani. Non soltanto gli addetti ai lavori, ma tutti gli italiani devono sapere che, grazie a questo lavoro di squadra, al quale tutto il Governo, a partire dalla sottoscritta, si è dedicato, ma che una volta tanto ci ha visto batterci, spalla a spalla, anche con esponenti delle opposizioni, abbiamo messo in sicurezza una percentuale significativa del nostro prodotto interno lordo, coniugando sostenibilità e competitività. Lo voglio citare, concludendo, come esempio virtuoso e come modello per il futuro perché quando l'Italia ha belle storie da raccontare, quando ha buone ragioni da difendere e, soprattutto, quando riesce a mettere l'interesse nazionale davanti agli interessi di parte,

il Presidente del Consiglio. Voglio salutare, a nome di tutta l'Assemblea, il Liceo scientifico «Augusto Righi» di Roma, che è venuto con i propri studenti e professori a farci visita.

un gesto - due dita e il pollice alzato puntati verso il Presidente del Consiglio - immediatamente represso da una delle insegnanti, che mi piace qui segnalare, per condannarlo nella maniera più decisiva, anche se posto in essere da un ragazzino.

*(FdI)*. Signor Presidente del Consiglio, ci troviamo oggi a discutere in vista di un Consiglio europeo particolarmente importante, perché gli scenari di guerra che si stanno prospettando all'orizzonte sono sempre più preoccupanti, la situazione in Ucraina, la guerra di Gaza e gli attacchi dei ribelli Houthi alla navigazione nel mar Rosso. Sono scenari foschi anche e soprattutto per le gravi difficoltà che stanno determinando e possono determinare per i commerci. Mi riferisco, in particolar modo, alla pericolosa *escalation* nel mar Rosso, dove la nostra missione Aspides dovrà svolgere il suo importantissimo compito, volto ad assicurare la sicurezza marittima, la libertà di navigazione, la salvaguardia del traffico delle merci. Ma non ci sarà pace nell'area senza che prima si riesca a dare una soluzione al rapporto tra Israele e Palestina. La risoluzione che andiamo ad approvare impegna il Governo a perseguire ogni sforzo per il raggiungimento, in prospettiva, di una soluzione di pace basata sulla formula dei due Stati, che vivono uno accanto all'altro, in pace e in reciproca sicurezza. Condividiamo quanto auspicato dal presidente Mattarella per l'Ucraina e il Medio Oriente. Queste guerre vanno fermate. sperando che il mondo possa tornare presto a sorridere. Come Italia dobbiamo proseguire, ancor di più adesso, come Presidenza di turno del G7, l'azione di mediazione alla ricerca di un negoziato giusto per il superamento delle crisi, con un intenso intenso impegno diplomatico per il raggiungimento di una pausa umanitaria a tutela delle popolazioni civili, fino ad arrivare ad un cessate il fuoco finalizzato anche a cancellare sangue e odio. Un tassello fondamentale del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo sarà l'agricoltura. È stato un merito particolare del Governo italiano, che lo ha fatto inserire all'ordine del giorno. Erano tanti anni che non veniva trattato in termini precisi il tema dell'agricoltura e, grazie all'azione del Governo Meloni e del ministro Lollobrigida, finalmente ci troviamo a discutere di questo. C'è una situazione di eccezionale gravità, perché è in corso una crisi di sistema a livello mondiale. La crisi geopolitica indotta dall'aggressione della Russia all'Ucraina, la crisi mediorientale, la chiusura parziale degli approvvigionamenti del canale di Suez sono tutti tasselli di una situazione drammatica che si riverbera direttamente sulle nostre produzioni. È importante, quindi, che l'Europa torni a parlare di agricoltura come prevedono i trattati europei, perché è una politica centrale per lo sviluppo economico della nostra Europa tesa alla sicurezza alimentare. D'altra parte, senza un'adeguata redditività per gli agricoltori, si spopolano le nostre campagne. Questo perché, nel tempo, la PAC ha visto sempre meno l'agricoltore come garante del territorio, ma piuttosto come soggetto in competizione con l'ambiente. Invece, in Europa noi abbiamo già chiesto, lo confermiamo anche oggi, un rafforzamento del ruolo dell'agricoltore. L'Italia ha chiesto anche la semplificazione dell'*iter* degli aiuti e l'estensione del periodo temporaneo di crisi, come avvenne per il Covid-19, per le imprese agricole in difficoltà. Inoltre, abbiamo chiesto che la normativa sulle pratiche sleali venga estesa a livello europeo. L'obiettivo per il nostro Paese resta quello di realizzare una PAC che favorisca l'agricoltura italiana, il lavoro dei nostri agricoltori, la qualità e l'unicità delle nostre produzioni. D'altra parte, già venerdì scorso la Commissione europea ha proposto modifiche che hanno l'obiettivo di alleggerire ulteriormente l'onere amministrativo per gli agricoltori dell'UE e di offrire agli agricoltori e agli Stati membri una maggiore flessibilità nel rispetto di alcune condizioni ambientali, senza ridurre il livello generale di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi ambientali e di protezione del clima della politica agricola dell'Unione europea. I nostri agricoltori si trovano ad affrontare crescenti incertezze, ma - grazie alle modifiche proposte - sarà possibile applicare alcuni *standard* in modo più compatibile con le realtà quotidiane che gli agricoltori devono affrontare sul campo. Dobbiamo difendere ciò per cui la Politica agricola comune è stata concepita sin dalle origini, vale a dire tutelare un reddito per gli agricoltori, che assicuri loro un tenore di vita ragionevole al pari dei redditi derivanti dagli altri settori produttivi. Gli agricoltori non solo provvedono alla produzione di cibo di qualità per tutta la popolazione, ma, al contempo, assicurano anche la tutela del territorio, la difesa dell'assetto idrogeologico e il mantenimento di un tessuto rurale vitale. Un'altra questione che sta a cuore al Governo Meloni è il tema dei flussi migratori e la loro gestione. Stiamo portando avanti il Piano Mattei. Dobbiamo lavorare con convinzione per dare concretezza ai sei pilastri del Piano, anche e soprattutto lavorando in sede europea sull'istruzione e formazione, sulla sanità, sull'acqua ed igiene, sull'agricoltura, sull'energia e sulle infrastrutture. La Presidente del Consiglio è stata in Egitto nei giorni scorsi anche per stipulare importanti accordi bilaterali *(Applausi)* riconducibili proprio alla realizzazione del Piano Mattei per l'Africa e per far fronte al flusso migratorio illegale contro i trafficanti di migranti. Particolare significato hanno anche i due Accordi di cooperazione firmati dal vice ministro Cirielli e, ancora, convenzioni finanziarie, intese e *memorandum*. Tanto è stato fatto. Infine, un ultimo punto a favore, anche se non è espressamente oggetto del Consiglio europeo - come ha detto il presidente Meloni - ci piace evidenziare. Tale punto riguarda la direttiva sugli imballaggi, su cui nei giorni scorsi c'è stato un importante accordo che ha raccolto le posizioni sostenute dall'Italia e anche da noi in Commissione affari europei, già nel 2022, all'inizio della legislatura, avevamo esaminato e criticato la proposta iniziale della Commissione europea. Abbiamo dimostrato che c'è un'Italia che non si arrende a soluzioni che penalizzano la nostra industria e che è capace di continuare a negoziare fino alla fine in maniera decisa, facendo valere la bontà dei propri argomenti, valorizzando le nostre eccellenze e riuscendo a modificare sostanzialmente il risultato. Ringraziamo quindi il *premier* Meloni che ha raggiunto importanti risultati, che sono però anche il frutto di uno sforzo corale di tutti gli attori del sistema. Siamo certi che il nostro *Leader*, cui rinnoviamo la nostra incondizionata fiducia, porterà in Europa ancora una volta un'Italia a testa alta, fiera e coraggiosa, pronta nuovamente a battersi per le proprie idee. Esprimo, in conclusione, solidarietà

riguarda l'Ucraina. Putin non si fermerà e non si fermerà perché non si è fermato. Kiev ha bisogno più che mai di sostegno, di armi e munizioni - lo dico anche alla mia parte - di una prospettiva certa, chiaroveggente perfino; di un'iniziativa europea che non sia solo di impulso americano, vista l'*impasse*

In Europa è il *Premier* ungherese a fare gli interessi di chi frena - usiamo un eufemismo sull'Ucraina - e qui da noi, nella vostra maggioranza, il lavoro di erosione lo fa la Lega. A poco vale dire, Presidente, che poi si vota tutti insieme, perché non c'è bisogno di aver studiato Austin per sapere che dire è fare; dire e disdire, Presidente Meloni, come si è visto ieri, e ieri, e i pannicelli delle smentite o delle rettifiche non coprono la vergogna - ripeto - la vergogna. *(Applausi)*. Le chiedo: è questo il basso continuo cui dobbiamo abituarci di qui a giugno? Mentre voi provate a rappattumare una posizione purché sia, l'Ucraina combatte sotto il fuoco incessante della Russia dove

Il senso di responsabilità la porterà a troncare, sopire, andare avanti e a fare finta che, ma sarà sempre peggio di qui a giugno. Lo dice la dinamica proporzionalistica del voto europeo. E questo è un problema non solo interno della maggioranza, ma è anche dell'Italia. Mi dirà: ma allora voi con il MoVimento 5 Stelle avete altrettante differenze sulla politica estera, non meno brucianti e per me dolorose assai. Giusto, ma, Presidente, noi non siamo il Governo del Paese, come voi, e ciò rende il nostro confronto - che c'è, che ci sarà, ed eccome se ci sarà - meno stringente oggi rispetto al vostro, meno urgente sul piano internazionale, su quello che si deve

presidente Meloni, di assicurarla a Bruxelles domani e nei prossimi mesi? Se denunciamo un'Europa recalcitrante, non possiamo essere altrettanto - se non più - reticenti. Se stigmatizziamo, come ella spesso fa, la cautela europea, non possiamo intiepidirci perché sennò la Lega ci chiede l'emendamento sul terzo mandato. Abbiamo già visto troppa campagna elettorale in Egitto, Presidente, Presidente, troppo silenzio: un nome e un cognome, quello di Giulio Regeni *(Applausi)*, che lei ha fatto qui oggi in quest'Aula, per pensare di poterlo tollerare nei mesi che verranno sull'Ucraina. In secondo luogo, Presidente, cito la Bielorussia. Il collega Terzi di Sant'Agata ha preparato un documento parlamentare che ho firmato: nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, si adoperi perché la sua maggioranza lo porti in Aula e lo voti per dare un segno udibile di quanto crediamo in una prospettiva di libertà in Bielorussia. Siamo il Paese nel mondo con il più nutrito gruppo di amicizia verso la Bielorussia libera e democratica. Si prodighi - la prego - perché non solo si sappia, ma si veda anche. Da ultimo, tutto questo impianto porta alla discussione sulla difesa europea, che è priorità assoluta. Più che sul fantomatico commissario alla difesa - con quali poteri poi vedremo - combatta per gli eurobond per finanziare i vari capitoli di bilancio prioritari: ambiente, innovazione, inclusione, ma anche difesa. Mi dirà che è la Germania a frenare, ma le rispondo che è esattamente in queste occasioni che si deve vedere l'autorevolezza di un Paese come il nostro. Se non si vuole lasciare spazio alla baldanza francese o alla sopraccigliosa prudenza tedesca, tocca all'Italia, tocca a lei fare la politica. Basta con un'Italia che serve solo a parlare con Orbán, campo di azione peraltro assai ristretto, visto che i sovranisti del PIS, suo partito alleato, sono stati per fortuna rispediti a casa dal voto. Non possiamo più farci bastare l'Ungheria, con buona pace di Petőfi e Lukács. Presidente. Eurobond subito per la difesa e per la pace europea. *(Applausi)*. *(FdI)*. Signor Presidente del Consiglio, Governo, onorevoli colleghi, finalmente torna l'economia al centro dell'agenda del Consiglio e lo fa su *input* del presidente Meloni, che pone sul piatto il tema più importante, quello dell'agricoltura in Italia e in Europa; argomento che era già centrale nei Trattati di Roma del 1957, ma sempre meno attenzionato nel corso del tempo dal punto di vista del reale sostegno. I nostri agricoltori attendono risposte: l'Europa deve darle e non perseguire nell'imporre vincoli assurdi ai prodotti e all'intera filiera produttiva come ha fatto sinora, depurandone la qualità e aprendo la strada alla concorrenza sleale dell'*italian sounding*. Imprese agricole, qualità, sicurezza alimentare devono essere i cardini sui quali implementare una reale politica agricola, come ha già dimostrato il lavoro costante e tenace del ministro Lollobrigida, improntato ad attenzione e concretezza. Puntando su questo, il Governo Meloni toglie il velo di Maya ad un argomento portato nel fondo della classifica delle priorità, riconoscendo finalmente che parlare di agricoltura vuol dire garantire sviluppo, ricchezza, benessere e tutela dell'ambiente non solo all'Italia, ma anche all'intero Continente. temi rilevanti sui quali bisogna investire con ogni strumento, in ogni settore, anche per superare il momento storico critico che ci vede attorniati da guerre. Il feroce attacco di Hamas del 7 ottobre ha riaperto scenari che non avremmo mai più voluto vedere e pone sul tavolo l'onerosa questione della tutela dei diritti umani in una terra dilaniata da un conflitto che dura da quasi un secolo. È importante perciò che la comunità internazionale introduca ogni opzione possibile, ogni sforzo necessario ad evitare ogni tipo di *escalation*. In quest'ottica, caro Presidente, va bene il *memorandum* di accordo con il Ministero della salute egiziano da lei annunciato per rafforzare la collaborazione nel campo degli aiuti umanitari ai civili feriti in arrivo da Gaza. Questo dimostra da parte sua una visione e un pragmatismo non scontati e conferma l'impegno ulteriore negli sforzi umanitari messi in campo dall'Italia fin dallo scoppio del conflitto. La crisi di Gaza deve raggiungere un cessate il fuoco, con la ferma convinzione che la sua definitiva soluzione non potrà che passare attraverso la creazione di due Stati. Alla possibilità di costruzione del processo di pace in Medio Oriente contribuirà sicuramente anche la pagina storica delle relazioni tra Egitto e Italia scritte nelle ultime ore con una serie di accordi bilaterali firmati al Cairo con il presidente al-Sisi nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa. Grazie all'impegno del Governo italiano, inoltre, anche l'Europa ha finalmente compreso che i flussi migratori vanno gestiti e non subiti e che con questo scopo è utile anche fare accordi con le Nazioni di origine e di transito degli immigrati per combattere i trafficanti di esseri umani. Lo stanziamento di 7,4 miliardi fino al 2027 per il *memorandum* fra Unione europea ed Egitto accompagnerà le sue riforme economiche e sociali, ma al contempo lo sosterrà per fronteggiare l'emergenza migranti. Come si vede, l'intuizione del Piano Mattei sblocca energie e collaborazioni nell'ottica di riscrivere il nostro futuro e quello dei partner nella direzione di lungo termine della stabilità sociale e politica, con buona pace, signor Presidente, di chi ritiene questi accordi insignificanti, vuoti o scandalosi e nasconde in questi aggettivi irresponsabili la contezza della sconfitta di decenni di politica di centrosinistra in questo campo inconcludente e demagogica. Nell'ambito del rafforzamento della sicurezza dell'Europa e in generale dell'Occidente si situa a pieno l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali. Il futuro dei Balcani occidentali è nella nostra Unione; la loro progressiva e graduale integrazione è fondamentale per costruire una base economica futura comune. futura comune. La loro inclusione serve al rafforzamento della sicurezza e allo sviluppo della resilienza comune. Come ha già dichiarato lei, signora Presidente del Consiglio, l'Europa ha una grande responsabilità verso i Balcani e deve impegnarsi per riaffermare il senso di appartenenza di questa regione al nostro mondo e ai nostri valori, senza contare che tutto questo porterà a rinnovare la presenza nelle nostre aziende in queste regioni e l'investimento nei settori strategici, con vantaggi reciproci, e l'avvio verso un mercato comune più solido e compatto. Infine, non bisogna trascurare la lotta contro la manipolazione delle informazioni da parte di soggetti stranieri e il miglioramento della cybersicurezza collettiva, due elementi essenziali delle guerre del ventunesimo secolo. Disinformazione, guerra ibrida, attacchi *hacker* ai principali siti istituzionali e di *asset* strategici sono, infatti, le nuove potenti armi con le quali confrontarsi ed è indispensabile avere sostegno e collaborazione da quanti più fronti possibili. L'importanza, poi, del supporto dell'Unione europea e dell'Italia nella difesa dell'Ucraina dall'aggressione russa è fondamentale, non solo per sostenere un Paese che sta lottando per la propria sovranità e integrità territoriale, ma per mantenere anche l'equilibrio geopolitico europeo, soprattutto per ribadire il principio di inviolabilità dei confini nazionali; un pilastro del diritto internazionale. Il sostegno italiano e dell'Unione europea si traduce in aiuti economici, umanitari e militari, dimostrando così un impegno concreto nella lotta contro un'aggressione ingiustificata e nel sostegno ai princìpi democratici. La *leadership* italiana, guidata dal nostro Presidente del Consiglio, si pone in prima linea nella promozione di un approccio europeo unitario e coeso di fronte a queste sfide. L'unità europea e la solidarietà tra gli Stati membri sono più cruciali che mai per affrontare con determinazione ed efficacia le minacce alla sicurezza internazionale e per promuovere la pace e la stabilità a livello globale. La nostra Nazione, forte del suo ruolo storico di ponte tra diverse culture e civiltà, può giocare un ruolo chiave in questo contesto, facendo leva sulla propria esperienza diplomatica e sulla capacità di mediare tra le parti.

Nell'esprimere piena solidarietà agli ucraini e a tutti i popoli che in questo momento sono sotto l'egida delle dittature, augurando un futuro di libertà e una nuova Patria per tutti costoro costruita sul valore della vita, ribadisco che noi italiani, noi europei, saremo sempre dalla parte dei diritti umani, della crescita e dello sviluppo dei popoli e della tutela delle libertà fondamentali di tutti.

quando si parla di riunioni ai vertici europei non posso non pensare alla mia esperienza di europarlamentare: un lavoro quotidiano per rappresentare al meglio gli interessi dell'Italia, dei nostri territori, affinché non si ripetano mai più periodi bui come quelli in cui Presidenti del Consiglio, che avrebbero dovuto rappresentare la nostra Nazione, si recavano a Bruxelles con il cappello in mano. Ricordo la supponenza di alcuni colleghi - ed erano quelli del campo largo che ci indicavano cosa fare e cosa non fare, con sguardi dall'alto in basso, grandi discorsi su una maggiore integrazione europea per poi vederli fare meramente i loro interessi. Purtroppo, a livello comunitario vediamo come spesso non vi siano interessi comuni e oserei dire nemmeno interessi diversi, ma addirittura opposti. Il dirigismo europeo per anni non ha visto nessuna opposizione del nostro Paese e ha fatto sì che i nostri cittadini e i nostri lavoratori subissero le conseguenze negative di anni di governi italiani che non difendevano gli interessi nazionali per paura di sfigurare in qualche bel salotto, al grido di «più Europa», danneggiavano la nostra economia, la nostra agricoltura e inserivano ulteriori vincoli burocratici e tasse per le nostre imprese. Ma come Lega e come Governo possiamo dire agli italiani che le cose stanno davvero cambiando. Tutto perfetto? Certamente no, no, molto evidentemente ancora deve essere fatto, ma possiamo rivendicare una postura italiana in Europa, da Padri fondatori e non da Paese che si accoda, o peggio si sottomette. Lo facciamo anche in politica estera, dove per la prima volta vediamo come Stati europei ci seguono e non siamo noi ad inseguire loro. L'abbiamo visto, signor Presidente, con l'accordo Italia-Albania, lo vediamo con il Piano Mattei e anche con i recenti accordi di cui lei ha parlato, siglati con Tunisia ed Egitto. Lo stiamo vedendo anche nei tentativi di trasformare il nostro Paese in un *hub* energetico, perché, cari colleghi, la sicurezza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico fondamentali per la ripresa dell'economia italiana e chi invece pensa che tutto debba diventare *green*, che tutti debbano andare con il monopattino e che le auto debbano essere tutte elettriche, non fa un dispetto al Governo o alla Lega, ma un grande regalo alla Cina. Sulla questione migratoria ci sono diversi *report* - lo ha indicato anche lei, presidente Meloni - che già segnalano un calo delle partenze dalla Tunisia grazie agli accordi siglati dal Governo. Molto di più evidentemente deve essere fatto, ma la strada è sicuramente quella giusta e sarà necessario guardare non solo ai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ma anche ai Paesi del Sahel, Niger su tutti, aree di partenza di questi migranti, per creare quelle condizioni - per citare un vecchio *slogan* della Lega - per aiutarli a casa loro, affinché abbiano il diritto a rimanere nella loro terra. Massima attenzione deve essere anche posta a livello europeo a quelle che sono le mire russe e le mire cinesi in quegli Stati. Non possiamo lasciare che questi attori ostili controllino quelle zone nevralgiche e usino i flussi migratori anche come arma ibrida, per destabilizzare il nostro Paese e l'intero Continente europeo. A proposito di arma ibrida, è necessario, Presidente, discutere a fondo delle minacce ibride che il nostro Paese e l'Occidente intero stanno anche in questi giorni subendo. Richiamo l'attenzione sull'ultimo *report* della nostra *intelligence*, a cui evidentemente va il nostro ringraziamento per l'importante lavoro svolto, sempre nell'ombra, in cui si segnala per la prima volta come la Cina, attraverso attività di penetrazione economica e altre ingerenze in campo sociale e culturale, ma anche accademico, abbia messo gli occhi sui nostri *asset* strategici nazionali. È fondamentale allora che il Governo ponga questa questione a Bruxelles, perché non riguarda solo il nostro Paese, ma anche altri *partner* europei, ed è necessario che anche la politica accenda su questo tema un faro. Da qui la mia richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta proprio sulle ingerenze straniere, affinché anche il Parlamento italiano possa discutere di questi temi fondamentali per la sicurezza nazionale. E guardate bene, lo fa proprio la Lega. Parlando di temi strategici, non posso non parlare dell'attuale difficile situazione internazionale. Sulla questione del mar Rosso, come Italia abbiamo avuto il coraggio di agire per primi e anche grazie alla nostra volonterosa e valorosa e valorosa Marina militare stiamo cercando di ristabilire la libertà di navigazione. Benissimo: un esempio concreto di come vadano difesi i nostri interessi nazionali. Proprio ricollegandomi alla questione del mar Rosso e dell'attivismo italiano, si è reso evidente come sia necessario avere una difesa, un Esercito, una Marina, un'Aeronautica capaci di intervenire ove e quando necessario. Gli investimenti in difesa si sono riscoperti cruciali e in questa direzione deve andare anche il nostro Paese. Vorrei poi aprire una riflessione su come coniugare al meglio gli aiuti per il sacrosanto diritto all'autodifesa del popolo ucraino con il mantenimento della strumentazione militare essenziale necessaria per la protezione territoriale del nostro Paese. La stessa riflessione si deve aprire anche sui tempi di rimpiazzamento degli armamenti che decidiamo di offrire: magari lavorare alacremente per completare la dotazione questi sono temi importantissimi e strategici per il nostro Paese e che a livello europeo devono essere discussi con la massima determinazione. potenziare le nostre capacità industriali di difesa, dando nuovo impulso anche al coordinamento con altri *partner* europei, ma occorre la massima cautela nel parlare di esercito europeo; più che di difesa europea, io parlerei di difesa dell'Europa, nell'ambito della quale gli Stati membri possono e devono fare la loro parte nell'ambito dell'Alleanza atlantica. Parlare di esercito europeo comune senza evidentemente una politica europea comune mi sembra un grave errore. Concludo con un riferimento a un punto della proposta di risoluzione che mi sta particolarmente a cuore. È una posizione chiara, netta, sancita anche dal ministro degli affari esteri Tajani e dal ministro della difesa Crosetto, ovverosia si esclude - l'ha detto anche lei, presidente Meloni, quest'oggi e qui noi siamo ad appoggiare questa tesi l'ipotesi dell'impiego diretto in operazioni belliche di contingenti militari italiani sul territorio ucraino. Qualcuno oltralpe parla di invio di truppe NATO e così facendo non solo mina l'unità dell'Occidente, che mai come in questo momento ha la necessità di rimanere unito, ma fa anche il gioco di Mosca e della sua *(Applausi)*. Ribadiamo il nostro posizionamento al fianco del popolo ucraino, un posizionamento saldamente ancorato ai valori occidentali, ma allo stesso tempo chiediamo di favorire ogni iniziativa diplomatica finalizzata ad una risoluzione del conflitto rispettosa evidentemente del diritto internazionale. Una missione che per impegno, serietà e responsabilità può e deve essere portata avanti da una grande Nazione come la nostra e da un Governo che ogni giorno si sta dimostrando sempre più all'altezza di questo difficile compito. Signor Presidente,

oggi in quest'Aula è risuonato il tema dell'agricoltura in più interventi, un tema molto sentito e di attualità di attualità non solo per le proteste in atto, ma perché coinvolge gran parte del territorio del nostro Paese. Con il massimo rispetto per il Governo in carica, per i Governi che lo sono stati e per quelli che lo saranno, riteniamo che il primato di mettere al centro l'agricoltura non l'abbiano i Governi, ma l'abbiano gli agricoltori, quelle donne e quegli uomini che nel dopoguerra si sono inventati un mestiere e che hanno fatto sì che tante aree interne del nostro Paese abbiano avuto quella valorizzazione produttiva che ci rende orgogliosi *(Applausi)* quando noi andiamo in giro per il mondo e vediamo negli scaffali dei supermercati, nei ristoranti e nelle enoteche i nostri prodotti, che sono figli di decenni e decenni di duro lavoro. Oggi ci dobbiamo tutti interrogare, se ci sono delle proteste; non si può solo scaricare sull'Europa, perché le politiche europee vanno di pari passo con le politiche nazionali. È in quel contesto che dobbiamo lavorare tutti per migliorare e per rendere più attuali e attuabili i bisogni del nostro sistema agricolo. Condividiamo e condivido il tema Meloni, ha sollevato in merito alla sburocratizzazione delle pratiche per l'accesso ai finanziamenti europei, ma ciò deve andare di pari passo con la sburocratizzazione delle pratiche anche in ambito nazionale e regionale. I nostri agricoltori passano troppo tempo a compilare moduli, libri, agende e lo sottraggono al lavoro delle loro aziende. Questo è un tema essenziale per la competitività delle imprese, così come lo è il giusto prezzo. Oggi è stato introdotto anche il suddetto tema alla fine della relazione, ma noi riteniamo che sia il punto principale: non ci può essere un'impresa se questa impresa non ha la sua redditività. Gli agricoltori non chiedono sussidi, essi chiedono di poter lavorare e di far sì che il loro prodotto sia remunerato per quello che vale, perché vale il sudore, come già detto, di tante donne e di tanti uomini. Ci dobbiamo interrogare sul perché non ci sia il giusto prezzo in agricoltura e dobbiamo pretendere a livello europeo provvedimenti che lo tutelino e lo garantiscano al pari della reciprocità che la Presidente oggi ci ha indicato e che anche noi condividiamo in tal senso. Un tema che non è risuonato in quest'Aula, ma che riteniamo fondamentale, è la formazione. Oggi il tema della manodopera in agricoltura è un grido d'allarme fortissimo. Dobbiamo pretendere e batterci perché anche i fondi europei sulla formazione in agricoltura siano messi a disposizione degli istituti tecnici e professionali agrari, per formare i nostri giovani verso un mestiere difficile

avvicinarsi a un mestiere estremamente complesso, anche per la sicurezza del loro operare in campo agricolo, che troppo spesso è considerata secondaria, il che non è accettabile in questa fase storica. In conclusione, abbiamo votato in quest'Aula un provvedimento sull'agricoltore come custode del territorio. Lo abbiamo votato perché ci crediamo, come crediamo che l'agricoltura e l'ambiente siano due facce della medesima medaglia: non esiste ambiente senza agricoltura, né agricoltura senza senza un agricoltore custode; per far sì che l'agricoltore sia protagonista di una giusta transizione, dobbiamo accompagnarlo e sostenerlo, ma soprattutto farlo lavorare in libertà.

so che quando un eminente professore dell'Università «La Sapienza» può inneggiare alla "compagna Luna", ci sono poi anche gli studentelli ignoranti che pensano di poter venire al Senato a mostrare il gesto Le vorrei dire, signor Presidente del Consiglio, che lei ha parlato più volte di orgoglio per gli obiettivi che ha raggiunto e per le cose che avete fatto lei e questo Governo.

e, quando lei si presentò in Parlamento per la prima volta come Presidente del Consiglio, ricordo l'*underdog*, il soffitto di vetro abbattuto e come come la guardassero dall'estero, ossia come una specie di marziano o un oggetto misterioso; ricordo anche che, prima di quelle elezioni, madame von der Leyen

Africa. Voglio ricordare che, in questi tempi così duri, l'Egitto è uno dei Paesi che si sta dimostrando migliore forse il Paese che sta svolgendo al meglio la sua missione di pacificatore, anche in termini di sostegno unitario nei confronti di ciò che accade a Gaza. Sono tutti aspetti sui quali riflettere. Ricordavo quante cose sono trascorse. Oggi le dico perché ha ragione a essere orgogliosa. Basta aprire «Il Sole 24 Ore la quota *record* da sempre: 34.000 punti; listino: più 60 per cento dal punto più basso ed era la metà di ottobre del 2022; imprese: più 477.000 assunzioni a marzo. Questo è il Paese

crescita in tutti i Paesi della UE: +3 per cento. Si tratta soprattutto di manifatture, di spesa delle famiglie, fondamentali e che aiutiamo, di turismo, che è un po' il nostro petrolio, di investimenti.

se proprio ieri, Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, perché di questo stiamo trattando, evocava un motto latino: *si vis pacem, para bellum*. qualcuno avrebbe fatto impressione, qualche tempo fa, eppure oggi è possibile dirlo, perché ci rendiamo conto di quali siano i tempi che stanno correndo.

verso la sicurezza collettiva, verso il progetto di difesa comune collettiva, il comune obiettivo della difesa europea, l'idea di progetti *dual use*, con impieghi tanto militari quanto civili, e i meccanismi di approvvigionamento. Inoltre, c'è

perché si assumano responsabilità comuni. È bello sventolare le bandiere della pace e gridare pace; dopodiché, bisogna rendersi conto di come funziona il mondo. A tale proposito lei, con fierezza, con orgoglio, con concretezza, ha fatto vedere un'Italia finalmente con la spina dorsale dritta. Sull'Ucraina, lei ha tenuto l'unica posizione possibile, quella giusta e doverosa. Non è

Non si può legittimare chi pensa o chi conta, attraverso la forza bruta o la minaccia delle armi, di cancellare un Paese e l'indipendenza di un Paese. La mia patria è dove si combatte la mia battaglia, dicevamo un tempo. È vero. *(Applausi)*. Senza di noi, non esisterebbe, oggi, questa Ucraina oggi, questa Ucraina libera. Voglio dire qualche cosa di più, anche se qualche anima candida magari si scandalizzerà. La pace non si fa alzando la bandiera bianca, anche se lo dice un Papa. Ma io ricordo un altro Papa, che diceva, invece, che la patria si difende in tutti i modi, anche imbracciando i fucili. Questo Papa è oggi santo. Era papa Giovanni Paolo II, che lo diceva per la sua Polonia, dimostrando all'Europa come si combatte con la forza della fede. non si fa nemmeno ipotizzando interventi militari per i pruriti muscolari di uno che, di solito, invero, si dimostra piuttosto femmineo. E capite di chi parlo.

Abbiamo dato l'esempio condannando senza se e senza ma gli aggressori, perché si sa qual è la parte aggredita e quale la parte degli aggressori, si sa chi sono i terroristi che hanno stuprato, che hanno rapito e ammazzato i bambini. Dopo di che non abbiamo rinunciato a riaffermare la posizione tradizionale italiana, che vuole la pace e vuole due popoli e due Stati, perché vuole la libertà e la giustizia per tutti. Gli interlocutori però, come ovvio, non possono essere quelli di un gruppo terrorista che prevede nel suo statuto l'eliminazione dello Stato di Israele. Siamo stati i primi a mandare la nave Vulcano. Sempre su scenari di guerra internazionali, stiamo guidando quella che è davvero la prima vera operazione di difesa europea. Sto parlando di Bab el-Mandeb, dove c'è la nave Caio Duilio, tra l'altro sottoposta a una pluralità di attacchi da parte degli Houthi. Stiamo difendendo non soltanto la circolazione e la navigazione internazionali, ma gli interessi primari dell'Italia.

con quel ruolo predatorio che è stato tipico di altri Paesi anche europei e che oggi è il ruolo che stanno giocando Russia e Cina. Signori, in Africa... *(Il microfono si *(FdI)*. Avrei voluto dire tante altre cose. Questo Governo ha saputo tutelare l'interesse nazionale, sa tutelare l'interesse nazionale, sa offrire l'immagine di un Paese che nel mondo difende la sua dignità, ma anche la libertà, la giustizia e il diritto internazionale. Dico quindi al Presidente Meloni di continuare così per davvero, con quell'orgoglio che ha rivendicato.

io in realtà non ho grandi difficoltà ad applaudire i colleghi della maggioranza. La linea sull'Ucraina e la linea su Israele, quelle che ci ha raccontato oggi la Presidente, sono corrette, se non che poi la maggioranza si si ricorda che per stare in quest'Aula o per fare politica ci vuole un certo tasso di virilità, mi pare di capire, come ha detto il collega Menia. tra dire cose giuste e poi, quando ci si distrae, ricordarsi che per fare politica bisogna essere virili, spiega le contraddizioni di questo Governo e spiega perché in politica estera è praticamente inaffidabile e poco credibile. credibile. La Presidente del Consiglio dice che loro parlano con tutti. Con tutti vuol dire con la Germania, la Francia, la Spagna e la Polonia, ma anche con Orbán. Capisce però anche un bambino che quando sei in una riunione di condominio, ci sono quelli che hanno molti millesimi e c'è il condomino che fa rumore di notte perché fa baccano nel condominio e nel cortile. Ora se tu ti accanisci a lavorare, non tanto con chi ha i millesimi, ma con chi fa baccano nel cortile, c'è il rischio che tu non riesca a portare a casa niente da quelle riunioni di condominio perché vieni accomunato a quello che fa baccano nel cortile. Stare dalla parte di Orbán e andare a dire in Ungheria «Dio, patria e famiglia», significa mettersi dalla parte di colui che vìola tutti i principi fondativi dell'Unione, significa perdere la propria credibilità. Così come si perde credibilità se si va a dire io sostengo Vox o il PIS, partiti che tra l'altro perdono le elezioni e i Governi che hanno vinto se lo ricordano. Allora il problema è che la politica estera del Governo, pur su contenuti condivisibili è molto debole. La sua debolezza si mostra, per esempio, quando il vice presidente del Consiglio Salvini, la cui assenza abbiamo tutti notato oggi, dice cose come quelle che ha detto sulla Russia. Quando dice che Navalny è morto e bisogna aspettare la fine delle indagini, fa per la prima volta manifestazione di garantismo, perché per Salvini non bisogna mai aspettare la fine delle indagini, si può andare subito in galera tranne per quanto riguarda la Russia. Quando Salvini dice che i russi comunque hanno votato, dimentica che in condizioni di vera democrazia avevano votato anche gli americani, eppure i sodali di Trump, che lui sostiene, hanno attaccato il Campidoglio e il popolo americano non aveva forse votato democraticamente per Biden? alla conclusione, perché purtroppo il tempo è tiranno. Se voi dite le cose giuste ma non fate le alleanze giuste perché siete poco credibili, succede che prendiamo sedici voti su Expo 2030,

il 13 dicembre alla Camera che non si fa politica con le fotografie, la verità è che noi abbiamo visto una foto con Scholz, Macron e Tusk, perché purtroppo quando c'è la politica estera, poi si fanno anche le fotografie.

Presidente Meloni, noi ci riconosciamo pienamente nella relazione e per questo ringraziamo ovviamente per la chiarezza e la franchezza. Sarà ancora una volta un Consiglio incentrato sulla risposta all'aggressione russa all'Ucraina, che invece bisogna continuare a sostenere finché sarà necessario, con l'obiettivo di consentire a Kiev di presentarsi poi al tavolo del negoziato quando arriverà il momento, per garantire una pace giusta nel rispetto della piena dignità dell'Ucraina e del suo coraggioso popolo. Ma per onore di verità, hanno stonato le ultime uscite del Presidente francese: non siamo favorevoli all'invio delle truppe, perché questo ci porterebbe a un'*escalation* del conflitto con esiti catastrofici. Il Presidente francese, forse per ragioni elettorali interne, per semplice eccesso di protagonismo, ha dato al mondo l'immagine di un'Europa divisa su tutto. Pensate che risate si è fatto Putin quando ha visto una foto a tre invece che a ventisette. Questo è il volto dell'Europa che non dovremmo mai mostrare perché la forza dell'Unione europea sta nella sua unità. Macron farebbe bene a imparare dalla storia recente, tornare indietro di qualche anno al giorno in cui Sarkozy lanciò l'offensiva alla Libia per abbattere Gheddafi. I danni di quella scelta li stiamo pagando tutti ancora oggi e proprio la Francia dovrebbe guardarsi bene dal ripetere gli errori del passato. Medio Oriente ribadiamo la nostra ferma condanna verso la brutale aggressione di Hamas contro Israele del 7 ottobre, lo dico con ancora più forza dopo aver visto con i miei occhi i resti del kibbutz e, permettetemi, abbiamo potuto vedere in questi giorni quanto siano state drammatiche le testimonianze degli stupri ai danni delle donne israeliane ed è stato davvero vergognoso vedere queste pseudo-femministe, nelle manifestazioni dell'8 marzo, espellere dai loro cortei donne come loro che chiedevano giustizia per altre donne colpevoli solo di essere israeliane. Detto questo, naturalmente nel nostro fermo sostegno al popolo di Israele, ribadiamo che la reazione di Israele deve avvenire nell'ambito della legalità internazionale, del diritto internazionale e umanitario e deve essere proporzionata. Per questo l'operazione di terra a Rafah è un errore; bisogna porre fine alla strage di civili innocenti, da una parte usati da Hamas come scudi umani per giustificare il mantenimento del potere corrotto e terrorista, dall'altra invece colpiti

È chiaro, dunque, che la cecità ideologica e la faziosità non portano da nessuna parte, non portano risultati, ma alimentano tensioni anche nelle piazze del nostro Paese. La crisi mediorientale, ovviamente, ha i suoi riflessi anche sulla questione del mar Rosso. A questo proposito, voglio unirmi alla gratitudine espressa alla Marina militare, all'equipaggio della nave Caio Duilio, impegnata nell'operazione Aspides guidata proprio dall'Italia, motivo di grande orgoglio e onore. I nostri marinai, che sono impegnati in quel tratto di mare per assicurare la libertà e la sicurezza della navigazione, sono elemento fondamentale per ripristinare i traffici commerciali, che devono essere assolutamente riattivati quanto prima per evitare l'aumento dei prezzi al consumo per le merci, legati all'allungamento delle rotte che tagliano fuori i porti mediterranei e segnatamente anche quelli italiani.

che finalmente l'Unione europea abbia sposato questa linea, fortemente sostenuta dall'Italia, di offrire di fatto un nuovo modello di cooperazione. È quindi fondamentale il coinvolgimento dell'Egitto nel controllo dei flussi migratori, con buona pace della sinistra, che non ha alcuna altra soluzione al problema migratorio che non sia la fallimentare ridistribuzione dei migranti, che non ha funzionato né nella sua forma volontaria, né in quella pseudo-obbligatoria per mancanza di volontà politica da parte di tutti gli Stati membri, compresi Francia e Germania.

questo Consiglio europeo si dibatterà anche di tematiche interne. È stato molto importante che l'Italia abbia chiesto e ottenuto una discussione specifica sull'agricoltura e non c'era bisogno del rombo dei trattori per sapere che il mondo agricolo sta fortemente soffrendo, soprattutto dopo la pandemia e dopo la guerra Di contro abbiamo avuto un appesantimento delle normative della burocrazia europea, soprattutto collegate alle normative *green* e tutto ciò va assolutamente rivisto. Per noi gli agricoltori sono fondamentali per la nostra sicurezza alimentare e per l'approvvigionamento di cibo di qualità, quindi dobbiamo sostenere questa categoria. bene la proposta della Commissione europea, che va finalmente nella giusta direzione. Noi crediamo che si possa fare ancora di più per semplificare l'eccesso di burocrazia ed essere così più coraggiosi anche nel dire una cosa fondamentale, cioè che non può esistere sicurezza alimentare, non può esistere agricoltura economicamente sostenibile se non c'è un approccio più pragmatico, meno ideologico alla transizione verde e se non si cambia l'approccio culturale nei confronti dell'agricoltore, che non è un nemico della natura e dell'ambiente rurale

Presidente del Consiglio, a ricordare il successo ottenuto sugli imballaggi: si partiva da una proposta molto penalizzante da parte della Commissione europea che non teneva assolutamente conto dell'eccellenza italiana, determinata anche da decenni di politiche sulla raccolta differenziata, di investimenti sulla tecnologia del riciclo. Ciò è stato in gran parte rivisto e sono state tutelate importantissime filiere industriali italiane.

del Consiglio, vada avanti così, è questo che deve fare un Governo politico dalle idee chiare, dai programmi precisi e coerenti con gli impegni presi con gli italiani. Mentre la sinistra resta ancorata a un passato non certo glorioso anche nei consessi europei, noi andiamo avanti per la nostra strada con la forza delle nostre idee, con grandi risultati che stiamo portando avanti, con un lavoro serio, attento, credibile

e, a distanza da più di due anni dalla brutale aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina, avremmo voluto ascoltare di un impegno finalmente concreto da parte del Governo, capace di imprimere un netto cambio di passo sul piano diplomatico. Purtroppo, infatti, nessuno intellettualmente onesto può negare che la strategia bellicista perseguita in questi due anni abbia fallito. ha fallito perché ha rafforzato Putin e l'economia russa, che è in forte espansione: il PIL russo ha registrato un +3,6 per cento nel 2023. Ha fallito perché ha indebolito la posizione militare e negoziale dell'Ucraina militare e negoziale dell'Ucraina e ha danneggiato l'Europa e l'Italia. Sappiamo bene quanto questa guerra è già costata ai cittadini italiani in termini di rincari delle bollette e in generale di notevole aumento del costo della vita. Solo gli Stati Uniti, oltre alla Russia, hanno guadagnato da questo conflitto, grazie alla vendita di armi e gas e il PIL degli Stati Uniti è cresciuto del 2,5 per cento signor Presidente, per suo tramite al Governo: chi vuole veramente difendere gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa e il benessere dei suoi cittadini deve lavorare per la pace e non per la guerra. Prolungare la guerra conviene a Putin, che, oltre ad avere una dotazione di armi e munizioni praticamente infinite, ha anche risorse umane praticamente infinite. Invece, fermare questo conflitto immediatamente conviene soprattutto all'Ucraina, che sarebbe ancora nella posizione di negoziare una pace e non una resa. Quindi, sempre per suo tramite, Presidente, esorto il Governo a trovare il coraggio di andare in Europa e sostenere con forza la via diplomatica quale unica via di uscita da questo conflitto *(Applausi)* questo Governo, leggendo testualmente le parole di papa Francesco, che nei giorni scorsi si è espresso dicendo che la parola «negoziare» è una parola coraggiosa: «Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna? Ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da mediatore». Oggi, per esempio, nella guerra in Ucraina, ci sono tanti che vogliono fare da mediatore. La Turchia si è offerta per questo e altri; non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore. Allora, presidente Meloni, sempre per suo tramite Presidente, ormai sei mesi fa aveva detto ai comici russi di avere delle idee per una via d'uscita dalla guerra accettabile da entrambe le parti e disse che aspettava il momento giusto per metterle sul tavolo. Ebbene, le do una notizia: è arrivato il momento giusto. Vada in Europa, si presenti a questo Consiglio europeo e abbia il coraggio di dare la sua soluzione e metta fine a questo conflitto russo-ucraino. Passiamo ora al conflitto israelo-palestinese e anche qui, colleghi e colleghe, Governo, vorrei sapere, sempre per suo tramite, presidente La Russa, se dopo 32.000 morti, di cui quasi la metà bambini, se dopo milioni di sfollati che stanno iniziando a morire di fame e che quando si mettono in fila per gli aiuti vengono presi di mira dai soldati israeliani, se c'è ancora qualcuno dentro quest'Aula che ha il coraggio di affermare che siamo di fronte ad un'operazione militare di autodifesa. Questa è una carneficina, è una punizione collettiva *(Applausi)* che vìola palesemente il diritto internazionale. Questa guerra va fermata ed è per questo che noi chiediamo un immediato cessate il fuoco, una missione ONU di interposizione e un processo di pace che vada di pari passo con il riconoscimento dello Stato di Palestina, perché va da sé che la soluzione di due Stati per due popoli presuppone che i palestinesi abbiano una loro entità statuale riconosciuta. Allora, anche qui, esorto il Governo e la presidente Meloni ad avere coraggio, a portare avanti in Europa l'impegno preso dal Governo rispetto alla mozione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza. Si tratta di una mozione fortemente voluta dalle opposizioni e passata solo con il voto delle opposizioni, perché la maggioranza - ricordiamolo ai cittadini che ci stanno ascoltando - si è astenuta. D'altronde, questo atteggiamento alla Ponzio Pilato è il medesimo tenuto dal Governo Meloni quando si è astenuto durante la votazione di ben due risoluzioni dell'ONU per il cessate il fuoco immediato. Coraggio, presidente Meloni, coraggio. La ricordo quando in più di un'occasione irrideva il presidente Conte assicurando che mai avrebbe avuto la sua postura nei consessi internazionali o in Europa. Europa. Per dimostrare al mondo intero il peso del nostro Paese nei rapporti con gli Stati Uniti, lei, presidente Meloni, che cosa ha fatto? Si è lasciata immortalare come la scolaretta diligente che riceve un bacio e una carezza per aver fatto bene i compiti a casa. Che statura, davvero impressionante. Che dire quando inveiva contro l'Europa e i poteri forti che mettevano in ginocchio il nostro Paese? Si è accorta, presidente Meloni, che mentre le banche festeggiano utili *record* pari a 28 miliardi grazie anche al rialzo dei tassi voluto dalla Banca centrale europea, in Italia, secondo il recente studio di Nomisma e di Save your home, due milioni di famiglie italiane rischiano di perdere la loro casa perché non riescono a pagare i mutui?

Infatti, Conte dall'Europa ha portato in Italia per tutti gli italiani 209 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lei, presidente Meloni, si è fatta assegnare con una telefonata, per il tramite del ministro Giorgetti, 12 miliardi l'anno di nuove tasse e nuovi tagli a sanità, istruzione, infrastrutture.

apre una nuova finestra") *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, *premier* Meloni, Ministri, Sottosegretari, colleghe senatrici e senatori, non so dove ci sta portando questa Europa; o meglio, lo so, ma non voglio pensar male, anche se le premesse ci sono tutte. Con l'adozione del *green new deal*, l'Unione europea sta mettendo a repentaglio interi settori produttivi in nome della sostenibilità ambientale. La formula legislativa della transizione verde, piena di incognite e sconnessa dal mondo reale, rappresenta un pericolo per milioni di lavoratori e rischia di distruggere l'economia europea così come la conosciamo La *nature restoration law* è una legge che, con il pretesto della tutela dell'ambiente, rischia di causare gravi danni all'agricoltura e agli agricoltori, i veri garanti del territorio. Questa Europa sta mettendo in campo politiche fallimentari che porteranno alla distruzione di intere filiere agroalimentari e all'esproprio di terre e campi ad uso agricolo, ad una nuova impennata dei prezzi per cittadini, famiglie ed imprese. Non solo i nostri agricoltori, ma quelli di tutta Europa si sono mobilitati nelle scorse settimane per manifestare contro queste politiche irresponsabili. Con l'approvazione di questa legge in nome dell'ideologia *green* da salotto, l'Unione europea corre verso il baratro consegnandoci nelle mani dei Paesi emergenti, *killer* dell'inquinamento mondiale e facendo perdere all'Italia la bellezza di circa 1.250.000 ettari attualmente coltivati, l'equivalente della superficie della Lombardia, con conseguente perdita di produttività e sicurezza alimentare; quella sicurezza che i nostri agricoltori garantiscono, a differenza di altri Paesi, anche europei. Mangiare italiano e produrre italiano è sinonimo di eccellenza, di qualità e di sicurezza alimentare, grazie ai nostri agricoltori e produttori. La Lega è da sempre al loro fianco. al nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, per fortuna l'Italia ci ha messo una pezza. Le follie *green* colpiscono anche il mondo industriale, in particolare la manifattura. Infatti dal 1° ottobre è entrato in vigore il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), considerato uno degli elementi chiave del "Fit for 55" e del *green deal*, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030, e di raggiungere nell'Unione europea la neutralità climatica nel 2050. Questo meccanismo è proprio un dazio ambientale, che chiunque importi tali materie prime - come appunto il cemento, l'energia e l'idrogeno sono classificati - deve pagare sicuramente.

dato che si troveranno a pagare un prezzo più alto per le merci, senza poter trasferire i maggiori costi sui prodotti finali, a causa della concorrenza dei prodotti finiti, importati da Paesi extraeuropei, con normative meno vincolanti. Non parliamo poi dell'accordo sulle case *green*: nonostante i correttivi apportati, il testo finale della direttiva rimane ancora oggi irrealizzabile in molti suoi aspetti, a cominciare dall'impatto stesso della normativa, contenente tutta una serie di obblighi e imposizioni legati al tema dell'efficientamento energetico, che avranno ricadute significative sui proprietari degli immobili. Le auto elettriche rappresentano uno dei punti di riferimento dell'integralismo *green*, anche se spesso si fanno i conti senza l'oste. La carenza di capacità della rete elettrica minaccia di diventare un problema non di poco conto sia per le famiglie sia per le imprese come ha dimostrato anche il *report* dell'olandese titolare dell'azione europea per il clima - che coinvolgerebbe 1,5 milioni di famiglie entro il 2030. Qualcuno a Bruxelles ha pensato bene a una direttiva che nel 2035 metta fuori mercato le auto a benzina e a diesel, a vantaggio del solo elettrico. Questa non è sostenibilità ambientale, ma il suicidio

Sul fronte migratorio non possiamo abbassare la guardia e pretendere sicuramente al più presto la firma dell'accordo sulla lotta ai trafficanti. L'Africa è strategica: noi non abbiamo materie prime, abbiamo bisogno di avere un rapporto costruttivo e non dobbiamo subire un'immigrazione che è terribile per le persone costrette a fare viaggi talvolta drammatici. Dobbiamo costruire professionalità e competenze per l'Africa, per aiutare quelle popolazioni a svilupparsi, come molti nostri missionari ci insegnano da anni, ma soprattutto come la Lega ha sempre detto: aiutiamoli a casa loro. Infine, presidente Meloni, quando finisce una guerra le testimonianze si riversano in varie forme e tra gli orrori emerge una nuova visione, quella del rinnovamento della speranza per un futuro migliore e di un mondo pacifista privo di guerre e bombardamenti, perché le generazioni future non debbano mai conoscere lo stesso destino. Perché dico questo? La guerra fra Russia e Ucraina si è piuttosto incancrenita, come pure la situazione tra Israele e Palestina. tramite il suo permesso, mi rivolgo alla *premier* Meloni affinché si faccia portavoce non solo di pace, ma anche di una richiesta di armistizio per fermare la strage di innocenti su tutti i territori.

perché la Terza guerra mondiale è l'ultima cosa che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli. Grazie, presidente Meloni, per la sua affermazione: vada in Europa e faccia valere i nostri interessi e i nostri valori, siamo al suo fianco. Mi associo ai colleghi per condannare il gesto fatto da quello studente verso di lei e verso le istituzioni e le esprimo la mia vicinanza.

questo ricordo dell'Aula. La tirannia dei tempi mi costringe ad essere brevissimo. Vorrei, allora, dire una cosa. Anzitutto, noi non esprimiamo gioia per l'esito delle elezioni russe. Non ci congratuliamo neanche con Putin e credo che sia assolutamente necessario stigmatizzare, ancora una volta, questo processo elettorale, che, se non fosse drammatico, sarebbe ridicolo, costruito sul sangue di Navalny. E bene farà il Consiglio europeo a chiedere la liberazione degli oppositori politici di Putin e a chiedere ancora l'applicazione di nuove sanzioni. vorrei dire alla collega del MoVimento 5 Stelle che ha appena parlato: per favore, non ridicolizziamo il tema dell'Ucraina. Non c'è stata una strategia bellicista. Colleghi, chi sarebbe l'interprete di questa strategia bellicista? Chi si è difeso? Zelensky sarebbe il bellicista? Noi che lo abbiamo aiutato? Forse dovremmo condannare l'unico bellicista vero, che è Putin, che è la Russia. *(Applausi)*. Perché sono loro che hanno violato il territorio dell'Ucraina e sono loro che hanno la chiave di ogni trattativa, che deve partire da un presupposto: il ritiro. E se non è possibile il ritiro, almeno l'istantanea fine dei combattimenti da parte dell'esercito russo. Allora si potrà intavolare una trattativa. Noi ci inchiniamo con rispetto a quanto ha detto il sommo Pontefice. Io non ho mai visto dei sommi pontefici, che interpretano la cristianità del mondo, che non abbiano espresso una richiesta di pace senza se e senza ma. È giusto che il Santo Padre abbia rivolto questa richiesta a tutte le autorità politiche e istituzionali, alle organizzazioni internazionali, che mai come oggi vedono drammaticamente diminuita la capacità di svolgere una qualche *moral suasion*. il multilateralismo è in una crisi drammatica, ragion per cui bisogna rifondarlo, non superarlo, perché non ci sono meccanismi diversi per concorrere alla vita della comunità internazionale.

possono fare proposte che noi non condividiamo, come io non condivido affatto la proposta estemporanea di Macron nei giorni scorsi, ma non mi sembra una buona ragione per mancargli di rispetto. *(Applausi)*. Bisogna resistere a sostenere l'Ucraina. La resistenza ucraina è assolutamente necessaria, se non vogliamo che il diritto internazionale venga messo sotto i piedi e vincano l'arroganza e la prevaricazione di chi ritiene che la forza militare possa essere l'elemento regolatorio del futuro. *(Applausi)*. Sui Balcani occidentali, sono assolutamente d'accordo con la strategia italiana. I Governi passano, ma i Balcani rimangono. Sono i nostri vicini e noi dobbiamo favorire il loro approdo in Europa. Se non facciamo questo, noi avremo sempre più rischi da quell'area del mondo. Pensate alle interferenze islamiche di tutti i tipi, alla criminalità che rischia di essere importata nel nostro Paese. Dunque, dobbiamo assicurare un futuro di stabilità europea a questa area del mondo. Noi siamo per dare una prospettiva europea ai nostri vicini e anche alla Bosnia Erzegovina, come ha detto prima, anche in Commissione esteri, il Ministro degli affari esteri. Medio Oriente dobbiamo parlarci chiaro e dobbiamo mettere le carte in tavola, senza ipocrisie. Sul Medio Oriente, signor Presidente, non c'è dubbio che quello del 7 ottobre sia stato un gesto hitleriano da parte di Hamas. Non c'è dubbio che nessuno di noi possa dimenticarlo. Non c'è dubbio anche che migliaia di palestinesi, a partire da bambini e donne, sono morti per questa reazione, a mio avviso, spropositata, a Gaza. Non c'è dubbio che noi in questi anni abbiamo tutti proclamato l'idea di due popoli, due Stati. Lei è stata solo recentemente al Governo, ma tante personalità politiche, in tutti questi anni, hanno sempre declamato lo *slogan* due popoli, due Stati. Vogliamo però dire la verità? Noi dicevamo due popoli, due Stati, poi gli insediamenti si moltiplicavano nel territorio della Cisgiordania e non abbiamo mai detto niente. Tutti noi abbiamo fatto finta di non capire che quegli insediamenti svuotavano qualsiasi presupposto di due popoli, due Stati. Israele è allora l'unica democrazia del Medio Oriente; è nel nostro codice genetico difendere Israele,

ma possiamo proclamare la nostra completa diversità. Netanyahu si è chiuso gli occhi quando arrivavano ingenti finanziamenti ad Hamas da parte dei Paesi del Golfo,

consentito ad Hamas una cosa drammatica, di impossessarsi cioè della questione palestinese. Noi sappiamo invece che Hamas non ha alcun interesse sulla questione palestinese *(Applausi)*, ma agisce per conto dell'Iran e forse, nell'equilibrio geopolitico mondiale,

Noi dobbiamo pensare però che le linee direttrici della politica estera americana sono molto meno distanti di quello che noi pensiamo.

di essere protagonisti di un'autodifesa che è fondamentale nel mondo e con le complessità geopolitiche che stiamo vivendo. Dobbiamo uscire quindi da una fase di minorità ed infantilismo politico istituzionale; l'Europa deve associare al polmone economico quello della politica estera e della difesa. *(Applausi)*. Questa è la battaglia italiana. Dopo di che, cari colleghi, c'è una certa discussione, che vede anche opinioni diverse, sul fatto se abbia fatto bene o meno il nostro Presidente del Consiglio a recarsi in Egitto. Io ho le mie opinioni, qualcuno ne ha altre. Io credo che i vicini non si scelgono, ma si trovano, e i nostri vicini sono la Tunisia, l'Algeria, la Libia, l'Egitto, il Libano e, in qualche modo, dobbiamo cercare di governare con loro un complesso Mediterraneo, dove il neo-ottomanesimo della Turchia sta diventando un *player* veramente significativo. Allora, colleghi, è il seguente: ha fatto bene il Presidente del Consiglio a richiamare il tema di Regeni perché non può essere una questione formale solamente per noi che facciamo politica convinti di certi valori. egiziano ha tutto l'interesse, proprio per implementare gli accordi che l'Unione europea sta facendo, a dimostrare serietà e la serietà si dimostra facilmente con degli indirizzi e dei dati anagrafici *(Applausi)* perché è l'unico modo per rendere protagonisti nel processo coloro che sono additati - poi si vedrà - come possibili colpevoli.

un senso di solidarietà commista a indignazione per il gesto di cui è stata oggetto. *(Applausi)*. Mi sono chiesto, nel sentire gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e ascoltando anche alcune frasi quasi di irrisione nei confronti dell'onorevole Presidente del Consiglio, se alla fine questi gesti non siano anche incoraggiati, purtroppo fra i più giovani, ma anche fra altri, da quello che talvolta si dice, dall'atteggiamento che si prende in quest'Aula nei confronti delle più alte cariche dello Stato, di cui sicuramente il Presidente del Consiglio della Repubblica italiana è l'espressione. Ringrazio con vivo apprezzamento il presidente Giorgia Meloni per la relazione, ulteriore conferma di un'azione di Governo sicura, concreta, incisiva, che dà la misura esatta di quanto la nostra Nazione sia diventata protagonista nell'Unione europea, protagonista con una maggioranza coesa nei voti e nei fatti, e lo dimostra la risoluzione di maggioranza che viene presentata su argomenti difficili dibattuti in tutto l'arco politico italiano e nell'opinione pubblica, sui temi che sono stati già affrontati: Medio Oriente, allargamento, Ucraina, sicurezza e difesa, agricoltura e immigrazione. Sull'Ucraina, la posizione del suo Governo, presidente Meloni, è assolutamente cristallina: garantiamo il sostegno dell'Unione europea a Kiev, sicuramente attraverso il Fondo di assistenza per l'Ucraina, ma anche ricorrendo a sanzioni più efficaci e possibilmente ai fondi russi congelati. È vitale anche mantenere l'attenzione a casi simbolici dell'attuale clima di violenza totalitaria che attraversa la Russia, con la morte di Navalny, la sua detenzione in condizioni disumane, le elezioni farsa totalmente prive dei requisiti minimi previsti dal diritto internazionale. È fondamentale ribadire la condanna per le azioni di Putin e per come egli stia trattando il suo stesso popolo. È importante sostenere attivamente Yulia Navalnaya, rappresentante di quella che è una vera Russia che vuole essere democratica e libera, la vera vincitrice morale delle elezioni farsa degli ultimi giorni. È lei che è stata la protagonista, con il suo coraggio e il coraggio di suo marito. Merita un sostegno concreto anche la presidente del Governo unitario di transizione per la Bielorussia, Sviatlana Tsikhanouskaya: dal 2020 la Tsikhanouskaya denuncia Lukashenko, che le ha sottratto la vittoria elettorale praticamente con un colpo di Stato e ha incarcerato o eliminato gli oppositori ed ora annulla persino passaporti e documenti per decine di migliaia di espatriati. L'Europa può e deve farsi sentire anche al Consiglio europeo. In questo senso va la risoluzione di maggioranza, perché c'è la necessità di provvedere all'estensione temporanea della validità dei passaporti e dei documenti dei bielorussi espatriati nell'Unione europea e probabilmente l'Unione europea può sostenere questi cittadini bielorussi nei modi opportuni e nelle forme nelle quali continuerà a sostenerli. Sorge naturale, parlando di tali crisi, il collegamento con l'industria della difesa europea: bisogna drasticamente accelerare l'acquisto di munizioni e materiali per Kiev e, se necessario, anche provvedendo a questo in Paesi terzi. Considerando, ad esempio, i cospicui interventi finanziari che abbiamo dovuto incontrare per superare la crisi del Covid-19, si deve pensare anche a una mutualizzazione di interventi a debito che possono essere molto cospicui, ma ci dobbiamo soprattutto rendere conto che le minacce alla sicurezza della nostra Nazione e dell'Unione europea sono altrettanto concrete e forse addirittura maggiori di quelle che abbiamo dovuto superare con la pandemia del Covid-19. Urge perciò attuare una strategia europea per l'industria della difesa in chiave di complementarietà con la NATO, con adeguate e ingenti risorse finanziarie. Questo concetto di complementarietà è stato ben presente nella sua relazione, onorevole Presidente del Consiglio, ed è sicuramente la strada da prendere. È nostro dovere e responsabilità, perché è in corso un vero e proprio attacco all'Europa. La scorsa settimana ho presieduto, alla presenza di altri colleghi,

che lei, signora Presidente del Consiglio, e l'onorevole Ministro degli affari esteri avete affrontato e ribadito come visione italiana precisa e operante in tutto quello che stiamo facendo. Sul Medio Oriente è certamente necessaria una continua, faticosa, forte azione di mediazione. Dal punto di vista degli interventi umanitari, ricordiamo l'intensa attività che sta svolgendo - è già stato detto - la nave ospedale Vulcano, che ha soccorso numerosi palestinesi, bambini feriti e malati e con loro i familiari che stanno arrivando in Italia. Il Governo Meloni è così in prima linea nel promuovere una soluzione di pace basata su due Stati che vivano uno accanto all'altro, in pace e reciproca sicurezza. Non dimentichiamoci questa frase fondamentale: deve essere tutta intera, così come tutto intero deve essere in riferimento all'articolo 11 della nostra Costituzione quando si parla di pace e di sicurezza. Condanniamo, fuori e dentro i nostri confini, i vergognosi episodi di intolleranza e violenza verificatisi dal 7 ottobre a questa parte e condanniamo fermamente ogni forma di antisemitismo: tolleranza zero per chi odia il popolo ebraico o demonizza lo Stato di Israele e la sua storia.

oltre che alla gestione dei flussi migratori, al Piano Mattei per l'Africa: un partenariato per lo sviluppo sostenibile che crea occupazione e promuove una cooperazione tra uguali, un decisivo punto di partenza con l'inaugurazione, avvenuta l'altro giorno, della cabina di regia presieduta dal presidente del ci rende orgogliosi del ruolo così eminente che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo Governo assicurano in Europa alla nostra Nazione.

che un gesto del genere, in un'Aula come questa, avvenga nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi. Anche io voglio unirmi a quello che il presidente Casini ha detto con un grande messaggio di vicinanza e di solidarietà alla famiglia di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, un servitore dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni. *(Applausi)*. Detto questo, io sarò molto breve, Presidente. Non ho moltissime cose da dire in replica, anche se ho trovato un dibattito sicuramente ricco di spunti, soprattutto ricco di molti elementi di condivisione, anche trasversali, in quest'Aula, che sono per me molto importanti. Chiaramente più è ampio il consenso che si può rappresentare sui grandi temi di politica internazionale, più l'Italia può presentarsi forte nei consessi nei quali Darò solamente qualche breve risposta su alcune cose che ho sentito, che invece non condivido, partendo dall'intervento del collega Filippo Sensi.

oltre alla linea politica che un Governo vota in Aula e rappresenta all'estero senza tentennamenti, che dimostri la compattezza di una maggioranza. E credo, senza timore di smentita e ringraziando le forze di maggioranza, che questo Governo in quest'anno e mezzo abbia sempre potuto rappresentare la stessa posizione con estrema forza e determinazione, come tutti a livello internazionale ci riconoscono e dispiace che spesso invece non venga riconosciuto a livello nazionale. Mi pare piuttosto che qualche tentennamento - mi consenta - ci sia dalle parti delle opposizioni e non faccio riferimento alla posizione del MoVimento 5 Stelle. Per una volta voglio fare riferimento alla posizione del Partito Democratico, perché è il suo partito che nell'ultima occasione si è astenuto, quando si è trattato di votare l'invio delle armi all'Ucraina. *(Applausi)*. Allora non si può avere due facce. Mi consenta, collega, non vale neanche dal mio punto di vista, l'argomentazione «vabbè, ma noi siamo all'opposizione, ci possiamo permettere di essere un po' *naïf*». Per carità, certo che non si hanno le stesse responsabilità di chi è al Governo, però io mi ricordo quando ero all'opposizione e penso che lo ricordi anche lei. *(Applausi)*. Penso che lei ricordi che Fratelli d'Italia ha tenuto, dall'opposizione, esattamente la stessa posizione che ha oggi che è al Governo, perché ci sono temi sui quali non si fa la campagna elettorale, per come la vedo io. *(Applausi)*. Ci sono temi che riguardano la dignità di una Nazione, che secondo me valgono un valgono un altro atteggiamento. Quindi, io che posso rivendicare un tempo nel quale lei ricorderà che c'era una maggioranza molto variegata al Governo di questa Nazione, se siamo onesti, ricorderemo che in un'occasione si era presentata da parte della maggioranza, che allora sosteneva il presidente Draghi, una risoluzione che io definii, nell'Aula della Camera, il manuale Cencelli della politica internazionale, nel senso che si tentava

chiara che alcune forze dell'allora maggioranza si astennero per consentire probabilmente al presidente Draghi di andare al Consiglio europeo con una posizione più chiara. Io l'ho sempre vista così. Dunque, penso che il problema da chiarire, sul quale vogliamo che sia la posizione italiana in tema di Ucraina, ad oggi stia più nell'opposizione che nella maggioranza. Sugli eurobond, sempre collega Sensi, per difesa e non soltanto, il Governo è d'accordo. Lei sa - ha già espresso questa posizione il ministro Tajani - che quando nella mia relazione parlavo di soluzioni e strumenti innovativi, mi riferivo soluzioni e strumenti innovativi, mi riferivo esattamente a questo. Così come sono d'accordo sul tema delle sanzioni sulla Bielorussia: c'è, come lei avrà visto, uno specifico paragrafo nella risoluzione di maggioranza. È molto chiara anche su questo e spero che vorrete sostenerla. Sulla vicenda del rapporto con Orbán, anche qui mi consenta di dire che non sono d'accordo, perché trattare come paria alcuni Paesi dell'Unione europea indebolisce l'Europa, non la rafforza. È esattamente quello che abbiamo visto e io trovo che, particolarmente in questo contesto, dividere l'Europa e indebolirla, per ragioni meramente politiche, ma di partito, sia irresponsabile. E sa perché, purtroppo, dico che sono ragioni politiche? Perché lei giustamente ha fatto riferimento (giustamente dal suo punto di vista) all'Ungheria. Qualche mese fa, collega Sensi, lei avrebbe fatto riferimento all'Ungheria e alla Polonia come le famose Nazioni di serie B, solo che adesso la Polonia ha cambiato Governo, in Polonia non c'è più un Governo conservatore e la Polonia da Paese di serie B è diventata un Paese di serie A.

prima erano Ungheria e Polonia; adesso è diventata l'Ungheria da sola, perché la Polonia ha cambiato Governo. Che cosa vuol dire? *(Commenti).* Significa banalmente che voi ritenete che vadano isolate le Nazioni che non hanno un Governo che considerate compatibile con le vostre idee Secondo me, particolarmente nell'attuale contesto, questa è una lettura di politica estera francamente sbagliata. Quindi, io opero diversamente ed è la ragione per la quale dialogo con tutti, anche con tantissimi *leader* dei quali non condivido la linea politica, certo. Quando devo fare gli interessi della mia Nazione, cerco di capire qual è l'interesse dell'interlocutore che ho di fronte. Per carità, ho i miei interessi di partito, sono fiera del mio partito, ma niente per me viene prima degli interessi che devo fare per la Nazione nel suo complesso. *(Applausi)*. Questa è la differenza fondamentale.

però che un giorno non le serva di dover ristrutturare tutto il condominio con i millesimi che ha anche il condomino antipatico; altrimenti temo che sarà tutto il condominio a pagare e non il condominio antipatico. È esattamente questo il problema. *(Applausi)*. Quando arrivano le decisioni importanti, chi le paga? Chi paga per l'isolamento di alcuni per ragioni politiche? Io la vedo così e penso che oggi l'Europa abbia ben altri problemi e debba riuscire a essere compatta, particolarmente in una fase come questa. E penso di averlo dimostrato, collega Scalfarotto. Se non fosse stato - diciamolo - per un importante impegno italiano; se non fosse stato grazie a una capacità di dialogo italiana, collega Scalfarotto; se non fosse stato grazie a quell'apertura e a quella capacità di dialogo italiana, lei oggi oggi non avrebbe la possibilità di continuare a sostenere l'Ucraina per i prossimi quattro anni. *(Applausi)*. Sono i risultati, a casa mia, che contano, e quei risultati li ha portati a casa la capacità di dialogo, e non il gioco a prendere il caffè con i nostri amici più importanti. Detto questo, ringrazio il collega

Confido che ci darete una mano, per le parole che lei ha espresso, nel dar loro le risposte che sono necessarie, a partire dal tema della sburocratizzazione anche a livello nazionale e regionale, che condivido e che condivido e raccolgo. Però anche qui mi si consenta, dobbiamo anche dirci le cose come stanno. Dobbiamo dirci che una discreta parte dei problemi che oggi gli agricoltori hanno dipende anche dalle politiche, dalle scelte ideologiche, in alcuni casi folli, che particolarmente la sinistra ha imposto in questi anni in Italia e in Europa. Ricordo ai colleghi, particolarmente a quelli del PD, che nel 2021 il PD presentò una mozione (Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut ed altri) per impegnare l'allora Governo «ad individuare una *road map* di uscita, entro un tempo determinato, dai sussidi ambientalmente dannosi che ne preveda la loro rimodulazione e/o eliminazione, a partire dalla prima iniziativa normativa utile». Fu una cosa sventata dal centrodestra. L'obiettivo era togliere i sussidi al gasolio agricolo. Al tempo non ci si riuscì. Questo Governo ha prorogato i sussidi sul gasolio agricolo, che è esattamente il problema per cui la gran parte degli agricoltori sta facendo contestazioni in tutta Europa. La giustificazione era sempre il *green deal*. La transizione ecologica - come abbiamo detto tante volte - deve poter correre di pari passo con la sostenibilità economica e ambientale, altrimenti rischiamo di andare dritti verso la deindustrializzazione. Collega Bevilacqua, alle iniziative concrete sul tema della pace - come ho detto - penso, per esempio, che le garanzie di sicurezza che noi abbiamo firmato e che voi avete contestato siano

mi si deve dire anche quali ne siano le condizioni. Sono mesi che chiedo al Movimento 5 Stelle di dirmi quali siano le condizioni che ritiene accettabili dal suo punto di vista: quando oggi si dice di negoziare una pace e non una resa - poi tornerò un attimo su questo punto - si ritiene, ad esempio, che la cessione dei territori attualmente occupati, in assenza di un ritiro delle truppe russe, sia un tema? Possiamo scendere tranquillamente nel concreto, ma il problema è che queste proposte

mi corre l'obbligo di ricordare che, quando Putin è entrato in Ucraina, per così dire, prevedeva una guerra lampo che sarebbe durata pochi giorni e avrebbe portato le truppe russe fino a Kiev, mentre oggi, dopo due anni, siamo in una situazione in cui l'ipotesi di un'invasione totale dell'Ucraina non è minimamente presa non è minimamente presa in considerazione su nessun *radar* e quella che le truppe ucraine arrivino a Kiev non è sul tappeto. L'Ucraina ha recuperato una serie di territori che erano stati occupati: questo, secondo me, non è un fallimento. Certo, se poi l'obiettivo era dire - come, in buona sostanza, si sostiene da tempo

se devo tenere per buone le parole che prende in considerazione, è perché qualcuno ha dato una mano all'Ucraina ad arrivare fin qui; se avessimo fatto quello che voi proponevate già diversi mesi fa, l'Ucraina si sarebbe banalmente arresa e sarebbe finita lì. Ovviamente, quanto al tema del costo del conflitto, i conflitti hanno sempre enormi difficoltà. Su questo voglio dire che, a maggior ragione perché l'Europa, nel suo complesso, affronta una situazione estremamente difficile sul piano economico, io penso che bisogna essere fieri dei risultati economici che l'Italia sta raccontando e che vengono raccontati da molti osservatori in queste settimane. Vale la pena ricordarne alcuni: *record* occupazionale; l'aumento del reddito medio delle famiglie; una delle due nazioni di tutti i Paesi OCSE nei quali aumenta il reddito reale delle famiglie. *(Commenti).* Capisco l'imbarazzo e capisco il nervosismo, colleghi. *(Applausi)*. Ancora, reddito medio delle famiglie che aumenta.

questi non sono numeri che ho inventato: sono numeri di organismi terzi. L'OCSE, un organismo terzo, dice che, nel 2023, i salari in Italia sono aumentati da tre a cinque volte tanto rispetto a quando al Governo c'eravate voi. Lo *spread* è ai minimi da due anni. Siamo il primo Paese in Europa nella realizzazione del PNRR. Nel 2023 l'Italia è cresciuta più della media europea. *(Applausi)*. Addirittura, l'Istat dice che è diminuito il rischio di povertà. Questo mi ha colpito, colleghi, perché io ero rimasta a quando la povertà l'avevamo abolita. Invece, se il rischio diminuisce, vuol dire che è ancora in vigore. La povertà è ancora in vigore.

PNRR, sentiamo ripetere, tutte le volte che veniamo in Aula, che, grazie alle capacità diplomatiche dell'allora Presidente del Consiglio, all'Italia è toccato il più alto ammontare di contributi del PNRR. Temo che non si sia mai letto

del Next Generation EU non veniva fatta in base a quanto fosse capace il Presidente del Consiglio. La distribuzione delle risorse del Next Generation EU veniva fatta in base a quanto fossero drammatici i parametri economici dei singoli Paesi. Quindi, la ragione per la quale l'Italia ha ricevuto l'ammontare più importante non è data dalle capacità diplomatiche dell'allora Governo, ma dal fatto che l'allora Governo avesse messo l'economia italiana in estrema difficoltà. Anche su questo bisogna fare un po' di storia: perché questa è storia, che vi piaccia oppure no.

Capisco la difficoltà. Ma anche qui continuo a sentir ripetere una cosa che non è corretta. In materia di Patto di stabilità, continuo a sentir ripetere che, con i vecchi parametri, noi avevamo la possibilità di fare il 3 per cento di *deficit*, mentre adesso, con i nuovi parametri, ci sarà la possibilità di fare l'1,5 per cento di *deficit*. Francamente mi stupisce, e mi preoccupa anche che qualcuno che è stato al Governo pensi

consentito un avanzo dello 0,25 per cento, al tempo. Quindi, con i nuovi parametri a regime, con la possibilità, anche per noi, di fare l'1,5 per cento di *deficit*, noi abbiamo una maggiore flessibilità dell'1,75 per cento rispetto ai vecchi parametri del Patto di stabilità. In miliardi, significa maggiore flessibilità per 35 miliardi. Forse si vuole fare demagogia. È politica, è il proprio lavoro e quindi si dicono delle cose che non sono vere. Ma io vi dico questo perché spero che non crediate davvero a quello che andate a raccontare in giro per l'Italia. Chi conosce un po' la materia si rende conto che, purtroppo, non si sa di che cosa

sulla lettura rispetto alla vicenda mediorientale, alla crisi di Gaza. Come lei probabilmente ricorderà, io ho detto dall'inizio degli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso che quell'aggressione così brutale, mostrata al mondo con quella disumanità, sembrava costruita quasi per costringere Israele a una reazione così forte da isolarla nel contesto internazionale. Sono passati mesi e sembra essere esattamente quello che sta accadendo sia nella Regione, sia a livello di opinioni pubbliche, anche da noi e in tutto l'Occidente. La ragione per la quale ritengo che oggi chi lavora per una *de-escalation*, per un cessate il fuoco almeno prolungato o chi lavora per dire - come io ho ribadito e ribadisco in ogni contesto - che dobbiamo lavorare concretamente da ora su una soluzione strutturale per il problema palestinese e, quindi, la soluzione due popoli, due Stati, lo fa soprattutto e anche nell'interesse di Israele. Questa è la linea che il Governo ha portato avanti fin dall'inizio e questa è la linea che, si spera, anche con il vostro sostegno, porteremo al prossimo Consiglio europeo. La ringrazio, Presidente, per essere stata attenta a tutto il dibattito e aver offerto attenzione a tutti gli interventi.

dalla mia Sicilia, Messina. Grazie agli studenti e ai professori.

parere favorevole sull'impegno n. 8 con la seguente riformulazione: espungere le parole da «esulando» fino a «della nostra comunità». Esprimo parere favorevole sugli impegni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9.

parere contrario sulle premesse e sugli impegni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e parere favorevole sull'impegno n.

e sugli impegni 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22 e 27. Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 1, con la seguente riformulazione: espungere le parole «rinnovato e più incisivo». parere favorevole sull'impegno n. 3, con la seguente riformulazione: espungere le parole «cessate il fuoco e il». Esprimo parere favorevole sull'impegno n. 4, con la seguente riformulazione: sostituire le parole «il rafforzamento» con le seguenti: «il pieno utilizzo». parere favorevole sull'impegno n. 7, con la seguente riformulazione: «a sostenere ogni iniziativa finalizzata ad accertare le circostanze della morte di Alexei Navalny». parere favorevole sull'impegno n. 9 con la seguente riformulazione: «a sostenere ogni eventuale iniziativa che favorisca il rilascio dei prigionieri politici, sia in Bielorussia che in Russia, nonché la fine delle persecuzioni delle opposizioni». parere favorevole: sull'impegno n. 10 con la seguente riformulazione: sostituire le parole: «immediato cessate il fuoco umanitario» con le seguenti: «una pausa umanitaria» ed espungere le parole da «continui» fino a «e senza restrizioni»;

«propri confini»; sull'impegno n. 28, con la seguente riformulazione: sostituire le parole da «nel processo di transizione ecologica» fino a «dell'ambiente» con le seguenti: «che garantiscano»; garantiscano»; sull'impegno 29, con la seguente riformulazione: espungere le parole da «alla realizzazione» fino a «coesione sociale». Esprimo infine parere favorevole sugli impegni nn. 2, 6, 8, 12, 17, 23, 24 e 25.

Signor Presidente, concentrerò il mio intervento sull'Ucraina, ma mi permetto di dare un consiglio alla Presidente del Consiglio. Su quella sedia ho visto tanti Presidenti prima di lei fare trionfalismo su dati economici e devo dire che non ha mai funzionato un granché, non ci sia qualche dato vero in quello che lei dice, ma perché per la famiglia italiana che ha difficoltà di accesso alle cure o di accesso al tempo pieno, è cambiato davvero molto poco. Le do un consiglio gratuito: eviti trionfalismi, perché l'opinione pubblica normalmente reagisce molto male. Io sono stato in Ucraina, come la Presidente del Consiglio, da poche settimane e vorrei che non ci nascondessimo qui il fatto che che la situazione in Ucraina è drammatica. E lo è per la semplice ragione che gli ucraini oggi sono in grado di sparare uno a sei

Secondo me, se fate un po' più di silenzio, quando parlo dei ragazzi morti in Ucraina, fate bene. Ma fate come vi pare. La riconversione economica russa è partita da parecchio tempo: oggi è in grado di produrre tre volte le munizioni dell'Occidente. Ma c'è un fatto che in queste settimane è avvenuto, ovvero le dichiarazioni di Putin e del suo collega Medvedev sono chiarissime: non c'è nessun desiderio di tregua. L'unica tregua possibile qui la può fare Santoro in televisione, quando va a un *talk show*. I russi non hanno alcuna intenzione di mollare e dunque noi dobbiamo chiamare le cose come si devono chiamare. Ci sono persone in quest'Aula che vogliono la resa dell'Ucraina e che contemporaneamente alzano un problema parlando di fascismo continuamente, quando qui il vero fascista si chiama Vladimir Putin, e questa dovrebbe essere una cosa trasversalmente riconosciuta. Il Congresso americano è paralizzato dai veti di Trump. I 5 miliardi di euro che l'Europa sta dando per le munizioni verrebbero utilizzati in pochissimi giorni, e uso il condizionale perché non stanno arrivando. Gli ucraini stanno tenendo Putin lontano da noi. Noi abbiamo 350 miliardi di euro di *asset* dei russi sequestrati, ma non li smobilitiamo. La verità è che le sanzioni occidentali sono ancora fatte da ridere: una parte consistente del missile ipersonico di Putin è costruita con componenti americane, e ancora accade. Noi non stiamo prendendo sul serio un un cambiamento della storia che ci mette di fronte a una Russia nuovamente aggressiva e che perdurerà per molto tempo a venire. Nonostante il presidente Macron sia un importante membro del Gruppo Renew, io non sono d'accordo con tutte e tre le cose che ha fatto in questo momento. In primo mandare (o dire che si vogliono mandare) soldati francesi senza coordinarlo in ambito NATO è un indebolimento del fronte europeo e rischia di aiutare Putin, piuttosto che danneggiarlo. In secondo luogo, le riunioni di condominio sono sbagliate. Chiunque tragga gioia dal vedere l'Italia esclusa da una riunione di grandi Paesi commette un gravissimo errore

tra gli applausi - mi spiace dirlo - non solo del Partito Democratico, ma di tutta la destra che non era al Governo, io dissi che quello era un insulto all'Italia e si sa che non ho particolare simpatia per il presidente Conte. Noi questo orgoglio dobbiamo ritrovarlo.

perché senza contenimento - come abbiamo fatto con l'Unione Sovietica - il rischio di una crisi è più ampio; in terzo luogo, non bisogna arrivare al conflitto diretto con la NATO. Questi sono i tre obiettivi che dobbiamo perseguire. Avendo detto questo, direi alla Presidente del Consiglio - se fosse qui - che ho anche apprezzato il suo intervento su Orbán quando c'era il rischio di veto sull'invio di armi in Ucraina. Ma non può sostenere

il Governo in senso astratto, ma l'appartenenza allo Stato di diritto, che è precisamente la ragione per cui noi sosteniamo gli ucraini contro un'autocrazia e una dittatura. Se la Presidente del Consiglio questo non lo ha chiaro, allora abbiamo un gravissimo problema.

è che gli unici campi di cui dovremmo parlare oggi sono divisi dall'atteggiamento nei confronti della crisi ucraina, della Russia e dell'estremismo. C'è in un campo chi vuole custodire i valori occidentali, chi sa che tutto ciò dipende dalla capacità di difendersi e quindi da un'Europa più unita,

e voi potete pensare che tutto questo possa essere messo sotto il tappeto? Forse è possibile farlo oggi, ma il confronto tra l'Occidente e le autocrazie aggressive, aggressive, tra chi è custode e applica valori democratici delle democrazie liberali e chi li vuole distruggere, andrà avanti per anni

Il suo Vice Presidente del Consiglio ha in essere un accordo con Russia Unita di Putin e non abbiamo mai visto una lettera di smentita. Giudica le elezioni russe della volontà del popolo, quando sappiamo che la democrazia liberale non è il processo di voto, ma è il processo di voto in un contesto libero. *(Applausi)*. E non è meglio Giuseppe Conte, che non dice niente, pensando che così non lo nota nessuno. Sono due facce dello stesso problema che destra e sinistra oggi hanno e che emergerà nel tempo. Non è più - scusatemi - il momento storico per cui si possa far finta di nulla, perché ci richiederanno di non far finta di nulla. E quando la guerra diventerà più difficile e il costo politico di sostenerla diventerà più ampio, lei vedrà, signora Presidente del Consiglio, quanto ci metterà il suo Vice Presidente a darsela a gambe. E voi vedrete quanto ci metterete, Partito Democratico, a incominciare a dire - avete già iniziato - che non si mandano armi, ma si manda materiale, come se fossero le muffole invernali e i Moon Boot. Questo è il punto, in cui noi dobbiamo sapere che il bipolarismo cadrà e dobbiamo prepararci, avendo chiaro che il campo non è largo, non è stretto, non è variopinto: chi difende l'Occidente, chi sta con l'Occidente, chi sta con l'Europa, perché solo sotto l'ombrello europeo siamo sicuri e chi non ha il coraggio di farlo. Chi non ha il coraggio di farlo non è un democratico vero.

Arriviamo ad oggi. All'attenzione di quest'Aula ci sono i lavori del prossimo Consiglio europeo, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo. Ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel corso del suo intervento ha ribadito la centralità assunta dall'Italia e ha rimarcato ancora una volta - semmai ce ne fosse bisogno - il profilo europeista dell'Esecutivo di questa maggioranza. Il prossimo Consiglio europeo si svolgerà praticamente a due mesi dalle elezioni europee del prossimo giugno, elezioni che rivestono un'importanza centrale per il futuro della nostra Europa. L'Europa, infatti, ha un impatto significativo sulle nostre scelte future, oggi sempre più influenzate dalle decisioni assunte in sede comunitaria. Sono convinto che l'Italia oggi, grazie a questo Governo, possa e debba far sentire forte la propria voce a Bruxelles, consapevoli che siamo uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea e che rappresentiamo dunque la storia di questa Europa. Nel prossimo Consiglio europeo si parlerà di diversi temi: difesa comune europea, Ucraina, agricoltura, migranti e, ancora, la crisi in Medio Oriente. Partiamo dall'Ucraina: non serve evidenziare in questa sede quanto sia essenziale e vitale non demordere nel sostegno nei confronti dell'Ucraina in questa guerra ingiusta e disumana. Abbiamo tutti in mente l'immagine del recente attacco a Odessa durante la visita del presidente Zelensky. Il pieno sostegno dell'Unione europea all'Ucraina e al suo popolo coraggioso non può e non deve assolutamente vacillare. Oggi più che mai è il momento che i 27 Paesi abbiano un'unica voce, forte e autorevole. Non servono fughe in avanti, ma c'è bisogno di unità e compattezza in Europa. Altro punto al centro dell'agenda sarà la difesa comune. Oggi più che mai nel contesto geopolitico attuale e nel quadro internazionale odierno, con la crisi in Medio Oriente e il conflitto in Ucraina, bisogna massimizzare gli sforzi per arrivare alla creazione di una difesa comune europea. Sicurezza e difesa sono fattori cruciali per il nostro futuro. Lo abbiamo visto con le scelte importanti fatte a protezione, ad esempio, del traffico mercantile nel mar Rosso e nel Golfo Persico, area nella quale transita il 40 per cento delle importazioni navali italiane. La missione europea Aspides, come è noto, è a guida operativa italiana. A tal proposito, un ringraziamento va alla Marina militare *(Applausi)* e all'equipaggio della nave Duilio, impegnata in una missione molto delicata e importante. La guida italiana dimostra quanto sia fondamentale la buona cooperazione fra tutti gli Stati dell'Unione europea. L'Europa è l'unico strumento che abbiamo per proteggerci. Da soli non andiamo da nessuna parte. Da soli rinunceremmo a giocare da protagonisti e lasceremmo la palla agli altri attori a livello globale, come la Russia, la Cina, gli Stati Uniti e molti altri. Ecco perché riteniamo che si debbano intensificare tutti gli sforzi per arrivare - come dicevo prima - a una difesa comune della nostra Europa. Sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare - lo abbiamo visto domenica scorsa con la sua missione in Egitto, presidente Meloni - l'Europa si muove nel solco tracciato proprio da lei. Sono partite le prime missioni operative in Africa del cosiddetto Piano Mattei. La cooperazione con i Paesi africani è la via giusta. Nove i Paesi coinvolti, sei le aree di intervento: sono questi i pilastri di un nuovo rapporto con l'Africa che - così come è avvenuto con la missione congiunta dell'Unione europea al Cairo e prima ancora in Tunisia, ad esempio - ha la finalità di arginare i flussi migratori irregolari. Rinsaldare i rapporti bilaterali italiani ed europei con il Presidente egiziano è cruciale, soprattutto in un momento in cui l'Egitto gioca un ruolo fondamentale anche sul fronte del conflitto in Medio Oriente, oltre che come Paese stabilizzatore geopolitico dell'area mediterranea. Sul tema dei migranti, dunque, prosegue la sintonia tra il Governo italiano e la Presidenza della Commissione europea. È una sintonia che rafforza il profilo europeista dell'Italia in questa fase storica. La crisi in Medio Oriente ancora oggi, a distanza di quasi sei mesi da quel 7 ottobre, è in cima alla nostra agenda. Purtroppo l'imperativo è trovare un linguaggio comune per condannare le violenze contro i civili da entrambe le parti, ma soprattutto per chiedere l'ingresso e la distribuzione in sicurezza di aiuti umanitari umanitari a Gaza. Va però garantito il rispetto e il diritto di Israele a difendersi. Ricordiamo infatti che è Hamas l'aggressore. Non possiamo accettare ambiguità: ogni forma di ambiguità su questi temi vuol dire lasciare spazi e rigurgiti di antisemitismo, che per noi sono inaccettabili. Va però garantita in parallelo la protezione dei civili, in linea con il diritto internazionale. In questo momento, sottoscriviamo le parole del presidente della Commissione UE von der Leyen: c'è solo un modo per ripristinare il flusso di aiuti umanitari ed è una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco. La situazione a Gaza, colleghi, è drammatica: bambini e anziani muoiono di fame. L'Europa, le cui radici cristiane rappresentano un pilastro valoriale non retorico ma autentico, ha il dovere di mobilitarsi a tutti i livelli affinché si trovi una soluzione adeguata. Tutti i percorsi devono essere utilizzati per raggiungere le persone che hanno disperato bisogno di aiuto. Altro tema del prossimo Consiglio europeo è l'agricoltura. Grazie al suo intervento, presidente Meloni, alla tenacia e all'impegno del ministro Lollobrigida, l'agricoltura dopo decenni torna ad essere centrale nell'agenda europea. Il Governo sta lavorando in queste ore a una revisione della politica agricola comune e anche al recepimento di alcune proposte italiane, come ad esempio la moratoria dei debiti delle nostre imprese agricole. È sacrosanto che a livello europeo ci sia la giusta attenzione a questo settore, rafforzando la politica agricola comune e individuando le risposte adeguate per contrastare la concorrenza sleale da parte di Paesi terzi. Presidente Meloni, come Italia chiediamo che gli aiuti alle imprese ci siano per coltivare e non per produrre di meno. Questo è uno degli aspetti fondamentali della storia Il mondo agricolo è una risorsa strategica; gli agricoltori sono i primi ambientalisti: a me piace definirli i migliori custodi dei nostri territori. L'agricoltura per noi è vita e non a caso lo chiamiamo settore primario, perché primario è il suo ruolo nella vita e nel tessuto sociale ed economico delle nostre comunità. I prossimi 21 e 22 marzo, l'Italia, grazie a questo Governo e a questa maggioranza, entrerà dalla porta principale del Consiglio europeo e non dalla porta di servizio, come in altre occasioni negli anni passati. Due settimane fa la missione del Governo negli Stati Uniti e in Canada ha rimarcato che l'Italia è saldamente ancorata al binario atlantista e a quello europeo, che si fondano sulla difesa della libertà, della democrazia e dei valori del mondo occidentale. Grazie a lei, presidente Meloni, l'Italia sta ricoprendo un ruolo importante e di grande prestigio a livello internazionale.

Grazie signora presidente Meloni, ho apprezzato gran parte del suo discorso, la sua fermezza senza zone d'ombra nel sostegno all'Ucraina e nella condanna della Russia, nonché sull'inaccettabile sproporzione della pur legittima reazione israeliana. Il mondo è cambiato e dobbiamo attrezzarci a viverlo per quello che è. Non basta più l'unione dei mercati e delle banche, ma occorre un salto di qualità nel processo d'integrazione tra gli Stati membri. Dobbiamo cambiare il processo decisionale con la maggioranza qualificata per quasi tutte le decisioni e dobbiamo investire molto di più per l'autonomia dei settori strategici, riducendo le nostre dipendenze dalla Russia e dalla Cina. Sulla difesa comune europea occorre giungere all'esercito europeo, da finanziare attraverso l'emissione di titoli di debito comune. Non possiamo essere erbivori in un mondo di carnivori, come ha giustamente detto il commissario Gentiloni. bene il suo impegno sull'Africa, ma i cinque miliardi del Piano Mattei sono una goccia rispetto al mare di risorse che manda la Cina. L'Europa per troppo tempo ha lasciato campo libero alla Russia su Paesi che fanno il bello e il cattivo tempo sui flussi migratori. E qui arrivo alle questioni che non mi convincono. Il fenomeno migratorio non può essere affrontato solo in termini emergenziali, visto che l'Italia ha molti più problemi con l'emigrazione dei propri giovani che con l'immigrazione dall'Africa. Tutte le proiezioni demografiche ed economiche dicono che abbiamo bisogno dei migranti, esattamente come dimostra il *click* *day* di ieri,

Ancor meno condivido la posizione di questo Governo sulla questione ambientale. Il *green new deal* è uno dei grandi meriti della Commissione europea di questi anni. Sebbene l'Italia sia uno dei Paesi più esposti ai cambiamenti climatici, cercate di frenare su tutto, dalle automobili alle case, dalle plastiche agli imballaggi, ma il vostro più grande terreno di scontro è l'agricoltura, in cui vi comportate da esecutori delle volontà delle *lobby* delle grandi aziende di pianura. Lo vediamo sulla difesa degli allevamenti intensivi, quando è ormai scientificamente dimostrato che sono una delle principali cause del cambiamento climatico, e lo fate dicendo che tutto deve restare com'è sempre stato, bollando ogni altra posizione come ideologica. Non si capisce poi cosa dovrebbe significare: forse l'ideologia di salvare il pianeta contro la vostra ideologia di soddisfare Coldiretti? Il colmo di questa vostra contorta filosofia lo avete raggiunto con il divieto della carne coltivata, quando la maggior parte degli altri Paesi investe in innovazione dalle grandi potenzialità. Siamo tutti d'accordo che bisogna tutelare i piccoli agricoltori, che sono i primi custodi dell'ambiente, ma le grandi fabbriche della carne non salvano alcunché, semmai inquinano e sono luoghi di grande sofferenza per gli animali, perché è di questo che stiamo parlando. allora di pensare al bene di tutti, non solo di una piccola fetta del vostro elettorato. Sulle questioni ambientali, serve un approccio molto più moderno e rivolto verso il futuro. Poi, nella sua narrazione c'è sempre troppo spirito nazionalistico. Invece, per costruire la casa comune europea serve soprattutto una grande rivoluzione culturale: non più gli italiani prima di tutti, i francesi prima di tutti, gli ungheresi prima di tutti, ma gli europei prima di tutti. Eliminate, allora, tutte le ambiguità che ancora ci sono nel vostro campo: l'alleanza con un antieuropeista e filoputiniano come Orbán o le inaccettabili prese di posizione del suo Vicepresidente del Consiglio, che paragona l'Europa alla droga per un tossicodipendente; per non dire delle sue affermazioni sulle libere elezioni in Russia. L'interesse e la credibilità del Governo di un Paese non possono in alcun modo essere sacrificate sull'altare di un presunto ritorno elettorale. Ora e dopo le elezioni europee abbiamo bisogno di un Governo che spinga l'Europa a farsi carico delle sue sfide.

prima del Consiglio europeo tutte le forze politiche danno sempre l'augurio di buon lavoro alla Presidente del Consiglio, perché rappresenta l'Italia. Noi non ci sottrarremo e, in uno spirito di bontà, abbiamo pure cercato di credere alle affermazioni che lei stava facendo. Mi spiace doverle dire, però, signora Presidente che, in un paio di passaggi, ella ha leggermente esagerato.

ma il dato al quale ella fa riferimento, quello del terzo trimestre del 2023, secondo i dati OCSE, è un dato drogato per un rimbalzo tecnico. La invito, invece, a guardare i dati Istat del quarto trimestre 2023, che segnano un -1.4

basta con questa sinistra europea che governa l'agricoltura. La presidente Meloni sicuramente sa che il Ministro dell'agricoltura italiano non si può definire di sinistra. La Presidente lo conosce bene,

il Commissario europeo per l'agricoltura si chiama Wojciechowski. Io ammetto di non averlo conosciuto prima: voi non so. Meloni lo dovrebbe conoscere, perché è iscritto al suo partito: è un polacco iscritto al suo partito in Europa.

uno sforzo di lealtà reciproco: lei non ci venga a raccontare barzellette in Aula e noi le rispondiamo con la politica. Il concetto di fondo, il primo punto, è il tema politico che pongo. Ursula von der Leyen Ursula von der Leyen è la Presidente della Commissione europea. Il nostro Gruppo europeo l'ha votata. L'hanno votata quelli di sinistra, l'hanno votata anche i grillini e l'ha votata Forza Italia. La Meloni non l'ha votata: onore al merito. Oggi, dopo cinque anni, io sostengo che Ursula von der Leyen sia stata un disastro: un disastro dal punto di vista ambientale, un disastro dal punto di vista istituzionale, un disastro dal punto di vista diplomatico. Invece, la Presidente del Consiglio oggi considera Ursula von der Leyen, un'interlocutrice, come è giusto che sia, ma una sorta di coperta di Linus per tutte le fotografie che deve fare. Quando infatti Salvini, cercando di fare a Pontida un'iniziativa con Marine Le Pen, anche in modo un po' provocatorio, fa un evento a Pontida - l'evento di Pontida - e la Meloni ospita Ursula von der Leyen a Lampedusa. Peraltro sui migranti segnalo, così per sicurezza nel caso facciano il *fact-checking*, 158.000 migranti arrivati nel 2023, 153.000 quando al Governo c'era quel

chiama in Emilia-Romagna; Bonaccini mi ha mandato un messaggio dicendomi che il miliardo e i 200 milioni ancora non l'hanno visto, aspettano un decreto del MEF. La Presidente chiama la von der Leyen in un'iniziativa diplomatica in Africa che noi giudichiamo anche con grande interesse, noi siamo favorevoli al Piano Mattei a livello teorico, se funziona.

e per quello che riguarda la nostra parte politica, siamo contrari a un nuovo mandato. Si può poi continuare a dire che non si fa politica con le foto, che vale per le foto con Biden o con Modi, bisogna però anche avere il coraggio di dire che nel 2016, dopo la Brexit, Italia, Francia e Germania si sono visti insieme a Ventotene. Nel 2022 Italia, Francia e Germania, dopo la guerra scatenata da Vladimir Putin, sono andate in treno a Kiev. Nel 2024 se al posto dell'Italia c'è la Polonia, io una domanda me la farei non perché godo nel fatto che non ci sia l'Italia, io esigo che ci sia l'Italia ed esigo che ci sia l'Italia perché penso che abbia una posizione importante da far sentire, con la civiltà di chi non viene in un'Aula del Parlamento a definire il Presidente della Repubblica francese un femmineo. *(Applausi)*. Questo dimostra la vostra incultura e la vostra mancanza di rispetto.

sarebbe servito anche a voi. Arrivo così rapidamente alla conclusione. Cara Presidente, diciamoci la verità, lei ha consapevolezza della difficoltà della sua squadra a livello internazionale. Non è un caso che, *unicum* negli ultimi anni, la Presidente del Consiglio abbia cambiato lo sherpa del G7. Voi direte che questi però sono argomenti poco importanti. No, cambiare lo sherpa del G7 a tre mesi dal G7 che si svolge in Italia, cioè a metà del lavoro, significa avere qualche problema interno. Del resto, basta vedere Instagram per capire che non c'è nessun hackeraggio ai danni dell'Italia, c'è qualche incapace a gestire i *social media* della Presidente del Consiglio. Così come non c'era nessuna aggressione russa quando un comico si spaccia per il presidente dell'Unione africana, è che qualcosa non funziona in quegli uffici. Allora, siccome io faccio il tifo perché l'Italia sia forte e credibile, sono contento che ci sia un cambio nella rotta, però mi domando perché si deve mettere alla guida dello sherpa del G7 la direttrice dei servizi segreti italiani. *(Applausi)*. Siccome io ho fatto la guerra perché quella signora non diventasse Presidente della Repubblica, perché penso che chi fa il capo dei servizi segreti deve fare il capo dei servizi segreti, sommessamente faccio notare che non c'è mai stato un direttore della CIA a fare lo sherpa del G7. C'è qualcosa che non funziona nel sistema istituzionale di questo Paese e non è un caso ciò che è successo su dossieropoli, nata da una denuncia del Ministro della difesa di questo Governo.

che però con questa storia non c'entra niente. Voglio dire, cara Presidente, che noi siamo dalla sua parte quando lei va in Europa, perché noi siamo per l'Italia. Quando però lei ha l'occasione di parlare al Parlamento, al di là delle battutine sulla destra e la sinistra, che è sempre colpa della sinistra, che ha rovinato tutto, persino sull'agricoltura quando governa la destra, ci faccia una cortesia signora Presidente, provi a sfidarci sulla politica. Noi concludiamo su questi tre temi che le poniamo. Il primo: noi diciamo che Ursula von der Leyen ha fallito, lei e il suo Governo siete in grado di avere una posizione unitaria su questo tema? *(Applausi)*. Le forze politiche di maggioranza hanno una posizione unitaria su questo tema? Il secondo: la Presidente ha fatto un grande lavoro su un tema e io voglio dargliene atto, perché Chico Forti tornerà a casa grazie all'azione diplomatica del Governo. *(Applausi)*. E siccome noi siamo intellettualmente onesti, riconosciamo che non era facile portarlo a casa, come era giusto portare a casa Silvia Baraldini, come è stato giusto portare a casa i marò, signora Presidente, lei ha il compito di portare a casa anche Ilaria Salis *(Applausi)* e lo deve fare dicendo agli ungheresi che se non rispettano lo Stato di diritto devono smettere di prendere i nostri soldi. ma finché qui non facciamo l'elezione diretta del Presidente della Commissione, saremo sempre nelle mani dei burocrati, perché l'Europa ha bisogno di un'unica grande riforma, ovvero il superamento del diritto di veto, l'elezione del Presidente della Commissione con elezione diretta e finalmente un percorso che ci porti agli Stati Uniti d'Europa. Noi ci siamo, non abbiamo capito dove siete voi.

con una intensità e con una drammaticità ancora maggiori di prima. Come è stato ricordato da tanti miei colleghi, stasera il Presidente della Repubblica francese ha parlato della possibilità di ingaggiare un conflitto mondiale inviando truppe della NATO a combattere contro la Russia lo ha fatto dopo averne discusso con il Cancelliere tedesco ed il *Premier* polacco. Il Presidente russo, a sua volta, ha minacciato di ricorrere alle armi nucleari. Si dice che sia soltanto propaganda elettorale, ma anche se fosse così, sarebbe una consolazione molto relativa. Se solo un paio d'anni fa un Capo di Stato avesse cercato di aumentare i propri consensi con questi argomenti, avrebbe evidentemente pagato un prezzo elettorale devastante. Come si vede, le cose sono cambiate radicalmente in brevissimo tempo. La guerra, quella guerra che la nostra Costituzione ripudia e che noi pensavamo fosse stata ripudiata dall'intera Europa, è tornata ad essere una presenza reale ed una minaccia incombente. La corsa al riarmo diventa la principale delle opzioni in campo. Noi per due anni, Presidente, siamo stati martellati da un paragone indebito: siamo tornati al 1939, c'è stato ripetuto ogni giorno, trattare con Putin vorrebbe dire cadere di nuovo nella funesta illusione di Monaco del 1938. io credo che i paragoni storici siano sempre discutibili, ma se volessimo rintracciare una qualche similitudine, questa sarebbe piuttosto con il 1914, quando l'Europa si avviò in perfetta incoscienza e forse senza che nessuno davvero lo volesse verso una tragedia inimmaginabile che in quel caso fu la Prima guerra mondiale. Il Ministro degli affari esteri italiano ha risposto alle ipotesi belliche avanzate in questi giorni vorrei dire con giusta fermezza e io non ho nessun imbarazzo a dire in questo caso che ci riconosciamo nelle sue parole. Ma questa posizione, pur giusta, non è affatto sufficiente. Non basta dire che siamo contrari all'*escalation,* di fatto alla guerra mondiale se poi non si fa nulla per fermare la slavina prima che questa ci travolga. L'Europa e l'Occidente non hanno mai cercato realmente una trattativa. Anche quando è stata nominata la necessità di un compromesso, lo si è fatto senza misurarsi con le condizioni reali. Una posizione secondo la quale è stato detto per mesi, per anni, che la guerra avrebbe dovuto continuare fino alla vittoria come è stata quella degli Stati Uniti e anche dell'Unione europea, di fatto non solo rende impossibile una trattativa, ma ha finito con il consolidare il potere di Putin. Ma come si fa a non vedere che trasformare una risposta all'aggressione in una crociata porta diritti alla terza guerra mondiale? Trattare significa invece cambiare strada, affermare una autonomia strategica nell'interesse di tutti e cominciare finalmente a svolgere un ruolo politico, quello che è completamente mancato in questi due anni e che ha reso la situazione di oggi ancora più complessa di prima. Servirebbe un segnale politico, un segnale che non equivalga ad una resa, anche perché più passa il tempo più quella dell'Ucraina rischia di diventare una resa sempre maggiore. Occorre un'assunzione di responsabilità: per cambiare strada bisogna smettere di inviare le armi. Un segnale del genere, una decisione coraggiosa assunta da un Paese importante e fondatore dell'Unione europea come l'Italia, avrebbe - questo sì - un significato non limitato alla sola guerra in Ucraina, ma avrebbe un'eco immediata nello stesso Medio Oriente, dove la reazione del tutto spropositata di Israele all'orrendo attacco terrorista di Hamas sta causando un massacro inaccettabile, una mattanza di civili che ripugna ad ogni coscienza civile e che deve essere fermata. La catastrofe umanitaria in corso a Gaza chiede il cessate il fuoco immediato. I bombardamenti sulla striscia, la privazione di elettricità, di cibo, di acqua sono un'intollerabile punizione collettiva che, secondo il diritto internazionale, equivale ad un crimine di guerra. Bisogna anche in questo caso prendere un'iniziativa. Io ricordo a quest'Assemblea che l'accordo di associazione tra Unione europea e Israele si basa sul principio guida del rispetto dei diritti umani. Questo significa che quell'accordo e i suoi princìpi fondanti vanno rispettati e che se questo non accade, se non si fermeranno gli attacchi sulla striscia, se non ci saranno chiare garanzie sulla cessazione della violazione dei diritti umani, allora quell'accordo va sospeso e vanno invece immaginate, di fronte al rifiuto di attuare il cessate il fuoco e di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite, misure sanzionatorie. Noi crediamo che, vista la situazione, si debba prendere in considerazione l'invio nella regione di una forza di interposizione, di osservazione internazionale e di supporto umanitario, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Per tutto questo serve un ruolo politico del nostro Paese, ma questo ruolo purtroppo non c'è. Si smetta di accettare le regole di un gioco suicida, come è stato finora; si provi a togliere la parola alle bombe, ai droni, agli eserciti, al riarmo; si restituisca un senso all'azione politica e soprattutto si restituisca all'Unione europea un'autonomia non solo politica ma strategica, che è l'unica condizione possibile per avere un protagonismo. Infine, vorrei fare un'ultima annotazione: ne hanno parlato in tanti e vorrei dire anch'io la mia sul suo recente viaggio in Egitto,

negando verità e giustizia per Giulio Regeni, significa esattamente tradire quella che vi piace tanto chiamare Nazione: vi dite patrioti, signora Presidente del Consiglio, ma su questo davvero avete umiliato l'Italia.

Signora Presidente, signora Presidente del Consiglio, colleghi senatori e membri del Governo, prima sentivo il senatore Renzi che ha parlato di varia umanità; pertanto, siccome si possono portare argomenti a piacere, credo che noi possiamo ricordare, come prima ha fatto la Presidente del Consiglio l'andamento della situazione economica che ci consente di affrontare l'Europa con un atteggiamento più determinato e forte di prima. Lo *spread* è sceso a 124 punti base ed è pari alla metà del valore massimo di 290 degli ultimi cinque anni; abbiamo avuto un record storico, ad esempio, per i BTP valore, con un collocamento record sui mercati di questi titoli pubblici, che sono comunque un indice dello stato di salute del Paese, quindi anche di chi lo governa. Il clima di fiducia dei consumatori aumenta, c'è un dato occupazionale positivo, con quasi 400.000 occupati in più nell'arco di dodici mesi; l'inflazione è tornata a livelli gestibili, non solo in Italia ma anche in altri Paesi. Quindi, abbiamo tanti fondamentali dati economici che non possono essere ignorati e questi ci consentono di affrontare il confronto e il dialogo europeo con maggiore forza e credibilità. Non a caso, l'abbiamo discusso anche nei giorni scorsi in questa stessa Aula con la presenza del ministro Fitto, le rate del PNRR vengono erogate, i soldi l'Italia li porta a casa, poi li dovrà utilizzare bene. L'ho ricordato e lo ribadisco: fa molto meglio l'Italia di quanto faccia, ad esempio, De Luca che fa i cortei a Roma, ma non usa i fondi europei in Campania. Sarebbe meglio che utilizzasse i fondi europei in Campania e facesse qualche corteo in meno Questa è la sinistra che non sa governare e non sa usare quei fondi. C'è il dato relativo all'immigrazione. Vedevo prima criticare gli accordi con l'Egitto e con la Tunisia, che noi rivendichiamo, perché non dimentichiamo l'esigenza di giustizia. In Italia è in corso un processo sulla vicenda Regeni, ma questo non ci impedisce di dialogare, in termini di *realpolitik*, con un Paese come l'Egitto che, voglio ricordare, contrasta il terrorismo fondamentalista, che ogni anno ha centinaia e centinaia di morti nelle sue Forze armate e nelle sue Forze di polizia, tragedia di cui non si parla, nel contrasto a un terrorismo fondamentalista che nel Sinai e altrove minaccia quel Paese. Se crollasse quella situazione, ci troveremmo degli altri Houthi - che già ci sono nel mar Rosso - forse anche sulle sponde del Mediterraneo. Troveremmo un altro contesto di crisi, come quelli che abbiamo nel Medio Oriente, nello Yemen, nel mar Rosso e ovviamente nella vicenda tragica di Gaza ed Israele. Abbiamo avuto dei risultati, anche negli accordi sull'immigrazione, perché a fronte di un'emergenza - perché tale è, nessuno l'ha mai negato - tra il 1° gennaio e il 17 marzo del 2024 c'è stata una diminuzione di circa 8.000 sbarchi. Sono stati rintracciati molti irregolari, c'è un primo effetto di questi accordi, perché noi stiamo facendo una politica politica umanitaria da un lato, con il Piano Mattei e gli aiuti a questi Paesi e, dall'altro, cerchiamo di bloccare l'attività dei mercanti di persone, che fanno un'attività che poi moltiplica le tragedie e le stragi nel Mediterraneo. Tutte cose che vengono discusse a livello europeo. Di Ucraina si è parlato molto oggi e vorrei dire anche al senatore Renzi che dà indicazioni a tutti: lui dice che non va bene la von der Leyen. Vedremo quello che accadrà, votano 27 Paesi. L'altra volta il Partito Popolare

Leyen. Non so se forse Renzi si distrae da queste vicende. Ho visto che dà ordini all'Europa il senatore Renzi. L'altro giorno ha detto che il presidente della Commissione doveva essere Draghi. Intanto, prenda il 4 per cento in Italia, poi darà ordini all'Europa. Faccia un programma per gradi. È un auspicio, perché vedo che già dice chi deve fare il Presidente della Commissione europea, ma io non mi preoccupo e neanche Draghi si preoccupa. Voglio dire che noi di Forza Italia faremo parte del primo Gruppo del Parlamento europeo e questa è una certezza, dopodiché gli altri vediamo se ci arrivano. Abbiamo tempo per verificare il tutto, tanto ci rivedremo in quest'Aula.

ha detto con chiarezza quello che pensiamo delle elezioni in Russia, la cui attendibilità è tendente allo zero, ma ha anche detto che l'Italia non è in guerra con la Russia. Attenzione, noi confermiamo il sostegno agli ucraini,

quando fa l'appello alla pace. Quando poi parla dell'ideologia *gender*, dell'aborto e di altre questioni, il Papa non viene citato, perché il Papa si cita quando usa alcuni argomenti e non in altre occasioni. Noi siamo stati chiari anche sul dire che non vogliamo un'*escalation* militare. Non vogliamo che la NATO entri in guerra con la Russia. Non vogliamo una terza guerra mondiale, ma non possiamo possiamo per questo abbandonare chi ha subìto un'aggressione. Vogliamo nel vertice europeo e in quelli che seguiranno porre i temi della difesa europea. La difesa europea è una priorità e un'emergenza, dobbiamo incrementare la nostra spesa per raggiungere i livelli previsti dalla NATO. Dobbiamo anche auspicare una maggiore collaborazione tra i Paesi e nella difesa, che può consentire poi un abbattimento delle spese. Sistemi d'arma, carri armati, armamenti: ci sono differenze tra vari Paesi europei; se ci fosse una convergenza, un programma comune, ci sarebbe anche un abbattimento di spese e una maggiore razionalizzazione. Quindi l'impegno per la difesa europea è fondamentale, è bene che l'Europa ne parli e noi siamo stati fautori del fatto che nel prossimo prossima Commissione, come detto anche dal Partito Popolare Europeo al recente Congresso di Bucarest, ci sia un commissario per la difesa per l'Europa, perché deve occuparsi di temi di questa natura. L'Italia potrà dire la sua: abbiamo non soltanto delle Forze armate che sanno farsi valere nelle missioni internazionali e abbiamo tutti elogiato oggi la nostra Marina. Ricordo - lo dico ai rappresentanti del Governo - che qualche giorno fa io alla Conferenza dei Capigruppo ironizzai perché qualcuno diceva di rinviare il dibattito sulla nave. Dissi: non è che gli Houthi aspettano il dibattito del Senato. Tirarono il

o delle emergenze fossero dettati dalle nostre riunioni e non invece, purtroppo, dalla follia fondamentalista degli Houthi che attaccano i liberi commerci nel mar Rosso, con tutte le conseguenze che ci possono essere. Sulla questione di Gaza, più volte il nostro Governo - e lo ha fatto il ministro degli esteri in particolare - ha detto che la ritorsione, l'intervento di Israele, ha superato limiti, che debbono anche essere comprensibili dopo quello che è accaduto il 7 ottobre. L'Italia ha svolto un ruolo importante anche di soccorso di bambini e di popolazioni, e vuole un impegno umanitario a Gaza. Tuttavia, dobbiamo ricordarci che quella del 7 ottobre è stata un'aggressione che, a mio avviso, ha fatto scattare nel popolo d'Israele e anche nelle comunità ebraiche nel mondo una sorta di sindrome dell'Olocausto. Infatti, un popolo che ha vissuto quella tragedia nel Novecento, quando ha visto all'alba di una giornata qualunque entrare nelle case della gente comune stupratori, violentatori e persone che hanno messo a fuoco i corpi di bambini, quella giornata credo che non la dimenticherà. La comunità internazionale deve ricordarsi che c'è stato un 7 ottobre; dopodiché dobbiamo fare tutti gli interventi necessari. Due popoli, due Due popoli, due Stati: certo, lo sappiamo, è una dottrina internazionale, un principio a cui il nostro Governo è anche vincolato. Però, mentre vedo due popoli, quello di Israele e il popolo palestinese, non vedo due Stati.

vedo il popolo palestinese, che si deve liberare dai terroristi di Hamas, che non sono uno Stato, ma una banda di assassini che portano guerra e tensioni nel mondo. *(Applausi)*. Questa è la realtà. Noi lo vogliamo uno Stato palestinese, ma uno Stato come quello di Israele, dove si vota, dove cambiano i Governi, dove c'è la Knesset, dove c'è dibattito. Invece non lo vediamo dall'altra parte, quindi ci auguriamo che sorga e che anche tra i palestinesi qualcuno faccia sentire la sua voce. Appoggiamo nel contesto del Consiglio europeo tutti gli impegni che il Governo ha annunciato anche oggi, che ha espresso con chiarezza e che nella proposta di risoluzione sono riassunti. Ma andiamo oltre la dimensione europea con la missione

per sentire una lezione diversa ora dall'uno e ora dall'altro. Il Governo ha mantenuto posizioni chiare nelle sedi internazionali, ha mantenuto posizioni che anche oggi la proposta di quindi andiamo avanti in questa strada. Non ignoriamo altri capitoli della materia europea, quell'argomento dei confini alla Bosnia Erzegovina e c'è il tema dell'Albania. Sono temi importanti e oggi è stato ricordato l'impegno sull'agricoltura che, per la prima volta, è stato è stato portato ai tavoli europei. Prendiamo poi un impegno importante e lo diciamo proprio noi di Forza Italia che, stando nel PPE, avremo sicuramente un ruolo centrale nella nuova politica europea che speriamo non sia condizionata dai socialisti, che tante cose sbagliate hanno imposto. Occorre riscrivere le direttive sulla casa, riscrivere le direttive sull'agricoltura, le direttive sull'auto, perché l'ambiente si deve difendere con indicazioni credibili, non con agende impossibili *(Applausi)* che scaricherebbero sulle tasche delle famiglie e delle imprese europee costi insostenibili. Il nostro è un europeismo attivo, da protagonisti e non da subalterni. Con questo spirito, quindi, noi votiamo ovviamente a favore della proposta di risoluzione che il nostro Gruppo ha contribuito a scrivere e diamo pieno sostegno al Governo, che in Europa si è fatto sentire e che anche in quelle missioni in Egitto e in Tunisia ha portato la Commissione europea, i Governi di altri Paesi e un'Italia protagonista e non subalterna. Questo oggi c'è e chi lo nega nega l'evidenza.

rimango sempre estremamente affascinato dalla dicotomia degli interventi del Presidente del Consiglio in quest'Aula: vedo cioè una Presidente che, quando prende la parola per le comunicazioni, legge il suo intervento con un *aplomb* istituzionale proprio del Presidente del Consiglio (poi, possiamo non essere d'accordo sulle cose che dice, ma le dice con quel rigore istituzionale che deve essere proprio di chi ha una così alta carica);

- cioè il vero Presidente del Consiglio, quella che dimostra di non avere alcun rispetto istituzionale per quest'Assemblea *(Applausi)*, a cui vuole dare lezioni su come si fa opposizione parla di tutto quello che non è stato fatto precedentemente, senza però dire cosa vuole fare questo Governo e ricordando invece soltanto quello che non è stato fatto. Le do una notizia, Presidente: fra dieci giorni, lei avrà governato più del presidente Draghi e più dei Governi Conte 2 e 1 *(Applausi)*, ma non abbiamo ancora capito nulla di quello che vuole fare per il Paese.

mangiata totalmente dall'inflazione: l'Istat con i dati del 2023 certifica un calo dell'1,2 per cento nel reale potere d'acquisto degli italiani.

ma piuttosto gente che non riesce a pagare il mutuo e due milioni di italiani che rischiano di perdere la casa. Questo è il quadro. Rispetto al Patto di stabilità,

in audizione ha detto che quel Patto di stabilità era il caos. Oggi lo festeggiate, buon per voi (e forse non per noi). Veniamo però ai temi del Consiglio quale si appresta a rappresentare il nostro Paese, Presidente. Nelle sue repliche ha ribaltato alcune questioni, a mio avviso, sul tema dell'Ucraina, perché ha detto che, nel momento in cui si decide di non proseguire nel sostegno militare all'Ucraina, si conferma il fatto che, se se avessimo iniziato il percorso in questo modo, avremmo visto l'invasione dell'Ucraina e ovviamente una resa immediata. Sta di fatto però che a oggi, dopo due anni, i territori occupati dalla Russia - illegittimamente, con la follia assassina di Putin, che va sempre ricordata - sono gli stessi che sono stati occupati dopo qualche settimana, a dimostrazione che il fallimento di questa strategia è legato allo stallo, che non è gratuito. È uno stallo che è costato 50.000 morti tra le truppe ucraine e 10.000 morti civili. Non sappiamo quante decine o forse centinaia di morti tra i militari russi, che sono esseri umani.

Lei ci chiede di chiarire la nostra posizione. Io mi chiedo, invece, che cosa intenda lei quando ha dichiarato testualmente, pochi minuti fa: come si può sedere ad un tavolo di trattativa con chi non ha mai rispettato gli accordi sottoscritti. È un principio sacrosanto. Putin non ha mai rispettato gli accordi. Ma se noi rifiutiamo l'idea di poterci sedere a un tavolo di trattativa,

avremo sconfitto la Russia: cosa che, purtroppo, potrà succedere solo passando per la terza guerra mondiale.

all'attentato terroristico terribile di Hamas, che è un'organizzazione terroristica. Ma io ritengo che si possa dire che già oggi quella proporzionalità non c'è più. Non c'è più, perché ci sono più di 30.000 morti civili, che non sono tutti militanti di Hamas. E oggi bisogna avere il coraggio di dire, con maggior vigore, che non si può accettare che ci sia una vendetta nei confronti del popolo palestinese.

Io non credo che, in prospettiva, quei bambini cresceranno con la volontà della pace e non con la volontà di vendicare la perdita dei loro genitori. Credo che ciò rappresenti per Israele, ma per il mondo intero, perché poi questi orfani diventano mine vaganti, che portano ad altri attentati terroristici. Quindi, oggi noi dobbiamo dire con più forza che non possiamo più accettare quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza e che vediamo quotidianamente. Le bombe che cadono su Gaza non proteggono Israele. Da quelle bombe nasceranno nuove tensioni, nuovi conflitti, nuova linfa per il terrorismo e non per la pace. Le ricadute ci sono anche per l'Europa, presidente Meloni. Basta vedere quello che succede nel Mar Rosso. Ci preoccupa anche la situazione in Cisgiordania, perché è evidente che c'è un allargamento degli insediamenti illegali, rispetto al quale, nel silenzio europeo, anche Washington ha assunto una posizione molto forte.

comune deve essere uno strumento e non il fine. Mi spiego meglio: alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, l'Europa ha deciso di unirsi dal punto di vista monetario, con un percorso molto lungo, che ha portato poi all'euro,

Siamo preoccupati dal pensiero che la strategia della politica di difesa comune diventi esclusivamente una questione industriale di produzione maggiore di armi e non sottenda invece l'esigenza di avere una politica estera comune *(Applausi)*, di cui la difesa comune è una parte. Senza una politica estera comune è molto più complicato pensare allo strumento di difesa comune. Tralascio il passaggio sull'immigrazione. Lei ha paragonato i dati 2023-2024, ha fatto bene. Se li paragoniamo a quelli del 2022, troviamo un altro *trend* di crescita e io credo che il 2023 sarà ricordato come l'anno *record* dell'immigrazione in questo Paese. Forse le ha portato un po' di sfortuna qualche titolo di giornale che diceva tam tam tra i migranti, c'è la Meloni non partiamo più. Ecco, poi son partiti ugualmente. *(Applausi)*. sul tema della politica agricola comune. In questi giorni mi sono trovato molto spesso a dover rispondere di campo largo, campo stretto, campo ampio; vorrei rispondere anche di campo agricolo in quest'Aula. Credo che sull'agricoltura italiana dobbiamo guardarci guardarci tutti negli occhi e dire che c'è bisogno di un sistema Paese che riconosca le necessità di un settore primario fondamentale per l'Italia, che deve essere tutelato, che ha un problema di sostenibilità del reddito enorme, che non è legato soltanto alle politiche europee, ma anche alla tipologia di mercato. Quello agricolo è l'unico imprenditore che non decide il prezzo di vendita dei suoi prodotti, li decide chi compra e già questo dimostra la fragilità di quel sistema. Dobbiamo lavorare assieme assieme come sistema Paese. Sono contento delle parole che lei ha usato rispetto alla PAC, a come è stata costruita e al momento in cui è nata. Sono parole di buon senso, come su questo tema sono sempre state quelle del ministro Lollobrigida che ringrazio. Credo che assieme dobbiamo chiedere le modifiche alla Politica agricola comune. Politica agricola comune. Quello che succede in Francia e in Germania, in particolare, avviene perché il piano strategico nazionale di quei due Paesi non è stato fatto nell'interesse collettivo degli agricoltori, ma in un modo in un modo approssimativo. Noi che abbiamo approvato il nostro piano strategico all'unanimità, in Conferenza Stato-Regioni e con delle risoluzioni di quest'Aula, abbiamo fatto un buon lavoro per tutelare i nostri agricoltori che di fatto in piazza ci vanno poco.

Signor Presidente, questo Consiglio europeo arriva in un momento storico in cui il mondo sta dando segnali molto preoccupanti. Sembra quasi un elenco della spesa, ma se andiamo a vedere cosa sta succedendo intorno a noi, siamo veramente molto preoccupati: la questione russo ucraina, di cui hanno parlato tutti i colleghi in quest'Aula; quella tra Israele e Hamas, di cui poi parleremo; le tensioni nel Golfo Persico; la Cina che ultimamente sulla questione con Taiwan continua a fare provocazioni per cercare di far capire chi è più forte; una preoccupante crescita dell'antisemitismo a livello europeo, ma anche nel nostro Paese e non dobbiamo voltare la faccia dall'altra parte. Senza contare le dichiarazioni del Papa e le dichiarazioni di Macron

al voto. È considerato un anno di grandissimi cambiamenti, tranne in Russia, dove abbiamo visto la situazione. In occasioni come queste il sistema Paese, Presidente, dovrebbe essere unito e coeso, far vedere al mondo, ai nostri connazionali e ai nostri concittadini che tutti noi stiamo dando una visione diversa rispetto al passato. Dovremmo dare una visione diversa rispetto al passato. che sta girando l'Europa e il mondo in modo autorevole, facendo capire che l'Italia non è quella che va con il piattino in mano a elemosinare.

il sogno di Gian Marco Centinaio. Una risoluzione unica di tutto il Parlamento *(Applausi)*, che dia al Presidente del Consiglio mandato per andare in Europa con un'Italia forte e con una politica forte che dica al Presidente del Consiglio: caro Presidente Meloni, tu rappresenti non la maggioranza, ma il sistema Paese. Sicuramente è il sogno di Gian Marco Centinaio *(Applausi)*, sicuramente non si avvererà mai, ma di dire che forse anche questa volta la politica un po' di debolezza la sta facendo vedere ai nostri concittadini. Presidente, noi abbiamo apprezzato moltissimo il suo intervento e glielo dico senza se e senza ma. Sulla questione russo-ucraina, lei ha parlato di pace giusta, ha utilizzato queste parole e l'abbiamo applaudita, perché ha parlato di pace, ma pace giusta vuol dire andare nella direzione che stiamo chiedendo noi. Quindi condividiamo il suo approccio, quello quello che c'è scritto nella risoluzione; condividiamo la condanna alla Russia, condividiamo il fatto che abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo l'Ucraina, ma

Mi spiace per i giovani studenti universitari, che dovrebbero studiare un po' di più prima di andare in giro con le bandiere della Palestina a dire che c'è una guerra tra Israele e la Palestina. C'è una guerra tra Israele e Hamas, perché noi il 7 ottobre non possiamo dimenticarlo. Il 7 ottobre abbiamo visto qualcuno che con un atto di forza ha creato una tragedia e ha dichiarato guerra perché Hamas nel suo DNA ha la soppressione dello Stato d'Israele *(Applausi)*. Non stiamo parlando, quindi, di una guerra israelo-palestinese, ma stiamo parlando di una guerra tra Israele e Hamas. Siamo d'accordo su quello che dice la Presidente, siamo d'accordo sul fatto che l'Italia e l'Europa debbano essere protagoniste in un percorso di pace e di aiuti umanitari, perché comunque in questo momento stanno pagando i tanti cittadini palestinesi tanti cittadini palestinesi per una guerra che non hanno voluto. Anche sotto questo punto di vista, quindi, è giusto che la presidente Meloni porti in Europa la voce dell'Italia. Anche sulla situazione del mar Rosso condividiamo le parole della Presidente e condividiamo il fatto che l'Italia sia protagonista il fatto che l'Italia sia protagonista nel Golfo. Questa è un'ottima cosa, semplicemente perché dobbiamo far sì che il Mediterraneo rimanga punto centrale dei trasporti delle merci e delle persone, perché dobbiamo far sì che l'Italia non diventi un posto di serie B, visto che se bloccano quel tratto di mare c'è da fare un percorso con le navi troppo lungo e il Mediterraneo sarebbe una rotta totalmente da dimenticare. Sul contrasto all'immigrazione clandestina, siamo dalla sua parte, Presidente, perché quando ci ha detto che l'Italia mette questa tematica sul tavolo tutte le volte che ci sono degli incontri al Consiglio, siamo dalla sua parte perché riteniamo che questa sia una tematica su cui l'Italia in più di un'occasione è stata abbandonata e lasciata da sola. Pensiamo - una risposta, tramite il nostro Presidente del Senato la voglio dare al collega Renzi - che giusto che la presidente Meloni parli con la presidente von der Leyen, perché è vero che la presidente Meloni è una *leader* di partito, ma è la nostra Presidente del Consiglio ed è giusto che abbia un'interlocuzione con la presidente von der Leyen. *(Applausi)*. Anche se noi abbiamo una posizione chiara e netta nei confronti di questa Europa, è giustissimo che lo Stato italiano parli con chi in questo momento sta governando - sicuramente male - l'Europa e dia buoni consigli,

un'ottima *mission*, perché dobbiamo andare in quella direzione e dobbiamo far sì che l'Africa diventi punto centrale e non sia ancora ancora una volta sfruttata da Cina e Russia. L'Africa deve essere aiutata a crescere, a evolversi, e sicuramente il ruolo del Piano Mattei, quello del nostro Paese e quello dell'Europa devono andare in questa direzione.

dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio si sono svegliati adesso, mentre questo Parlamento lo ha votato mesi fa. Per noi l'agricoltore custode del territorio è nel nostro DNA, ma se l'Europa si sveglia adesso, ben venga, cara Europa.

che la PAC debba rimanere invariata per l'Italia. Diversamente, se l'ampliamento a Est prevede meno soldi per gli agricoltori italiani, con gli agricoltori dell'Est Europa che oggi ci stanno facendo concorrenza sleale, allora non ci stiamo.

con il Governo italiano di fronte ad alcune questioni inerenti l'Ucraina, la sicurezza e la difesa, l'allargamento dell'Unione europea, il contesto sempre più complesso del Medio Oriente, le relazioni esterne, la migrazione, l'agricoltura e il semestre europeo. Devo confessarle che ai colleghi del Gruppo, che ringrazio (il senatore Casini, il senatore Franceschelli e il senatore Sensi), avevamo chiesto proprio una sintesi delle proposte del Partito Democratico per avere da lei un punto di vista chiaro su proposte

ci si risponda su quali sarebbero le divisioni all'interno del Partito Democratico, come se foste attenti ad un possibile nostro congresso o al rapporto tra noi e il MoVimento 5 Stelle o tra noi e il terzo polo. Signora Presidente del Consiglio, vorremmo parlare della posizione del Governo italiano nel Consiglio europeo e abbiamo bisogno di risposte. Siccome ci preoccupiamo della condizione italiana, le chiedo formalmente di dirci che cosa pensa delle parole del vice presidente del Consiglio Salvini *(Applausi)*, perché quelle parole offendono tutto il Paese Non è tema del Consiglio europeo, presidente Meloni, ma è tema da politica estera della Repubblica italiana *(Applausi)*, perché se un Vice Presidente dice una cosa e l'altro ne dice un'altra, mi chiedo come fa a non farsi una domanda: perché nel vertice contestato, che non ha fatto piacere nemmeno a noi, lo ha ribadito il senatore Casini prima, quello, per intenderci, tra Francia, Germania e Polonia, Polonia, non era stata avvertita? Perché in quei passaggi l'Italia non è stata nemmeno considerata, essendo l'Italia un punto fermo, cuore e cervello di questa Europa? Non ci ha fatto piacere, signora Presidente. Nelle sedi europee sono state costantemente ribadite alcune questioni, dalla ferma condanna all'aggressione russa all'Ucraina, che non abbiamo sentito dalla Lega, al pieno sostegno dell'Unione europea per tutto il tempo necessario al diritto naturale di autotutela - voglio ricordarlo soprattutto al collega Romeo in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite: il diritto internazionale per la sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale. Voglio essere chiaro: la posizione del Partito Democratico è cristallina e non consentiamo a nessuno di fare propaganda su questo. Se questa è la posizione europea, signora Presidente, vorremmo capire perché in questi giorni il Governo è sembrato più attento a giustificare le proprie posizioni in Europa, le posizioni diverse tra le forze politiche della maggioranza in Europa, anziché provare a rispondere ad alcune questioni. Sa perché glielo dico, signora Presidente,? Io non ho molto apprezzato il fatto che la Presidente del Consiglio, probabilmente

Se un partito politico, in un contesto, pone un tema di come affrontare la transizione ecologica e voi lo trasformate in una clava da abbattere contro una idea di

le parole del senatore Menia sono le parole del Gruppo Fratelli d'Italia. Mi piacerebbe sapere se sono le parole della maggioranza, mi piacerebbe sapere se questa visione dell'Europa, sempre e comunque considerata un nemico, sono le stesse, signora Presidente, che non io, non la segretaria o un collega del Partito Democratico, ma che lei, signora Presidente, citava sulla Russia nel 2015, sull'Europa nel 2016 e sulla Brexit del 2016, sull'euro del 2014 e del 2017. Signora Presidente, non gliele leggerò le sue dichiarazioni. Sa perché non gliele leggero? Perché, Perché, nonostante tutto, lei oggi fa la Presidente del Consiglio della Repubblica italiana e queste parole io penso lei le abbia rinnegate. Queste parole offendono la nostra idea di Europa: da «l'Italia dovrebbe assolutamente ritirare la sua firma, le sanzioni sono una cosa idiota per l'economia italiana» tra Obama e Putin «scelgo assolutamente Putin, credo che in politica internazionale Obama sia il peggiore Presidente degli Stati Uniti». Da allora in poi è stato un susseguirsi, e lei mi porta qui l'onorevole Pezzopane? Ma me ne porti tante di onorevoli Pezzopane *(Applausi)*, perché c'è la storia di un modo di concepire l'Europa rispetto alla quale non ci siete ancora.

il Patto di stabilità, rispetto al quale lei ci ha trascinato, sia migliore di quello originario; lo ha detto anche qui. Nonostante l'impegno del commissario Gentiloni, che aveva proposto una mediazione molto alta, lei ha trascinato l'Italia oltre i tempi supplementari. Ci ritroveremo l'anno prossimo oltre i tempi supplementari perché l'accordo fatto, come lei sa, è al ribasso rispetto alla proposta originaria fatta dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. *(Applausi)*. Il costo lo pagheremo noi; ripeto, Presidente Meloni, non sia nervosa, ascolti l'opposizione. Signor Presidente, da qualche parte dobbiamo provare a confrontarci, visto che nel merito non si entra mai. Siccome la presidente Meloni ha detto che l'accordo fatto in Italia è migliore rispetto al vecchio Patto di stabilità, tra l'altro sospeso e che noi non avremmo mai voluto rivedere, dico che, a causa dell'atteggiamento del ministro Giorgetti, che per mesi ha rinviato e ha buttato la palla in tribuna perché dentro dentro la maggioranza c'era una divisione profonda tra Lega e Fratelli d'Italia, il risultato è che abbiamo portato il nostro Paese ad una mediazione al ribasso. Quella mediazione, signora Presidente del Consiglio, la pagheremo e sa perché? Perché partiremo già da meno 15 miliardi, che sono le clausole che avete firmato, quelle del cuneo fiscale che sono a tempo determinato e quelle della pseudoriforma fiscale, perché per la prima volta nella storia il nostro Paese ha fatto una riforma fiscale solo per un anno. Quando però dovremo rinnovare cuneo

Signor Presidente, mi consenta di terminare. La Presidente del Consiglio ha parlato di condominio. Per dieci anni all'opposizione nel nostro Paese ha...

cosa fare e diamo, attraverso i suoi senatori, giudizi sui *leader* di altri Paesi con i quali noi non andiamo spesso d'accordo, ma c'è un rispetto istituzionale che abbiamo il dovere di mantenere. Concludo, signor Presidente, ribadendo un concetto. Per questa destra ancora nazionalista e antieuropea l'Europa non è un soggetto politico: non c'è un popolo europeo, non c'è una difesa comune possibile, non c'è un bilancio comune, non c'è un *welfare* comune. Non è; per questa maggioranza l'Europa semplicemente non è. Nonostante tutto, gli italiani l'8 e il 9 giugno dimostreranno che l'Europa è. *(Applausi. l'ultimo intervento, vediamo se lo riusciamo a fare senza disturbi e in tempo utile.

Signor presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, desidero innanzi tutto manifestare la solidarietà di tutto il Gruppo Fratelli d'Italia - che abbiamo apprezzato sia venuta anche da altri Gruppi - per il gesto che c'è stato da parte di uno studente. Ho avuto adesso la notizia dal senatore questore Nastri che la preside della scuola interessata ha già scritto una lettera scusandosi e spero che anche lo studente autore del gesto capisca che, se vuole difendere qualche idea, deve fare

neanche per un giorno, nei dieci mesi precedenti a questo Governo lo *spread* è stato così basso. Ci sono oltre 600.000 posti di lavoro in più, in gran parte stabili. C'è l'inflazione: se ne parlava tutti i giorni, quando era alta;

fondamentali che ne erano alla base sono effettivamente migliorati. Il fatto è che all'epoca l'11,8 per cento era ben al di sopra della media dell'Unione europea; oggi lo 0,8 di inflazione che c'è in Italia è il più basso tasso tra tutti i Paesi del G7 e in Europa è il più basso di tutti tranne di quello della Danimarca, che ha un'inflazione lievemente inferiore. Vorrei pertanto che si parlasse anche di questo, che tocca la vita quotidiana di tutti i cittadini, in particolare di coloro che hanno un reddito basso. Contemporaneamente, c'è stato un *record* di recupero dell'evasione fiscale e la Borsa proprio oggi ha superato il 62 per cento di guadagno rispetto a quando il Governo è entrato in carica. È aumentato il potere d'acquisto delle famiglie e il debito pubblico, esattamente in direzione contraria a quanto autorevoli esponenti della sinistra prevedevano prima delle elezioni, è sceso

*dossier* internazionali dà i suoi frutti anche sui due drammatici conflitti cui stiamo purtroppo stiamo assistendo. Questa posizione è quella giusta. La fermezza che è stata messa in atto rispetto al sostegno all'Ucraina, tenendo sempre presente chi è l'aggredito e chi è l'aggressore, rappresenta la posizione giusta: non servono le fughe in avanti, tantomeno quelle all'indietro. Con questa posizione si aprono le prospettive per avere un punto di riferimento certo nell'Italia e, per quanto sta all'Italia, anche in tutta l'Europa. La stessa questione riguarda la crisi di Gaza. Non dimentichiamo l'attacco del 7 ottobre: molti lo dimenticano. Non dimentichiamo che la stessa Hamas ha detto che vogliono farne il più possibile di questi attacchi, fino ad arrivare all'eliminazione dello Stato d'Israele. Lì sì, allora, che si parla di genocidio. Come ha detto la senatrice Segre, la parola genocidio è stata

Anche qui la posizione dell'Italia è stata estremamente chiara, dialogando con coloro con cui si può dialogare, cercando di fare il possibile per creare le condizioni per una pace nell'immediato e anche per una pace stabile nel futuro. Eppure l'opposizione non risparmia le critiche su tutto. In particolare, ho sentito, anche oggi, che si rimprovera a lei, signor Presidente del Consiglio,

che vengono in particolare dal Partito Democratico, non siano una sotterranea critica all'allora presidente del Consiglio Conte, che nel novembre del 2018 incontrò al-Sisi. Anche lui parlò del caso Regeni, ma senza ottenere nulla di diverso in questo senso. Il risultato diverso ottenuto da questo Governo è avere ottenuto la liberazione di Zaki. Non si dovrebbe poi parlare neppure con il Presidente tunisino, che peraltro è l'unico sostanziale esito duraturo delle famose primavere arabe varato dal presidente presidente Obama. Non bisognerebbe parlare con Saied. Non bisognerebbe parlare con la maggior parte dei governanti europei, perché bisogna parlare solo con il *club* di serie A, come lei ha detto, presidente Meloni. Io ricordo ai colleghi che la Germania, da sempre, parla proprio con quei Paesi coi quali si vorrebbe che l'Italia non parlasse, ancora prima che entrassero nell'Unione europea, con dei contatti intensi, attraverso le fondazioni dei vari partiti del centrodestra, di destra, della sinistra e del centro, creando quei rapporti che adesso stanno migliorando, grazie proprio al fatto che il presidente Meloni e questo Governo, in generale, parlano Grazie a questa interlocuzione, parlando con tutti, si sono ottenuti importanti risultati, dei quali io sono costretto a fare solo l'elenco. Sulla questione imballaggi, come lei ha ricordato, presidente

la proposta fatta da Gentiloni non è stata certamente bloccata dal Governo italiano, ma è stata bloccata dal Governo tedesco a guida socialista. Dunque, non possiamo dar la colpa al Governo Meloni di quello che è stato fatto da altri. *(Applausi)*. Se naturalmente l'ideale era fare esattamente ciò che volevamo noi, io ricordo che l'alternativa reale era tra il vecchio Patto di stabilità e quello attuale, che dà molta più flessibilità, in particolare all'Italia. E oltre a dare più flessibilità all'Italia, è più orientato agli investimenti, perché abbiamo visto che l'*austerity* e la riduzione di ogni tipo di intervento non hanno portato bene; anzi, hanno fatto aumentare il debito da parte di quelli che lo dovevano risanare. Io ricordo anche, tra i successi del Governo, il vertice Italia-Africa. Proprio in quest'Aula, poche settimane fa, c'erano decine di Capi di Governo e di Capi di Stato africani. Se ci fosse stata una politica più attenta negli scorsi decenni, non soltanto da parte dell'Italia, ma da parte dell'Unione europea

come patrioti, abbiamo il dovere e l'onore di darle il nostro pieno sostegno e, ringraziandola per aver detto di essere fiera ed orgogliosa del suo partito, diciamo che siamo molto fieri e molto orgogliosi di darle il nostro costante sostegno.

Ho il piacere di leggervi una lettera firmata dal dirigente scolastico, professoressa Cinzia Giacomobono del Liceo scientifico «Augusto Righi», che si riferisce all'episodio avvenuto nel corso della nostra seduta: «Signor Presidente del Senato, signora Presidente del Consiglio, questore anziano, ho appreso dalle insegnanti del gravissimo episodio avvenuto oggi durante la visita in Senato di una classe dell'Istituto da me diretto. Come corpo docente siamo colpiti e addolorati dall'episodio, che contrasta con il nostro impegno quotidiano per trasmettere ai ragazzi i valori del dialogo,

come noi. Mi scuso insieme ai docenti, accompagnatori e ai ragazzi per quanto accaduto che costituirà occasione di un approfondimento nel consiglio di classe e di una riflessione con i ragazzi. Vi prego di estendere le nostre scuse a tutta l'Aula del Senato e a tutto il Consiglio dei ministri. A nome delle docenti accompagnatrici, mi permetto

Spezzo una lancia affinché non ci sia un'eccessiva punizione, essendo già sufficiente quello che abbiamo visto qui.

È stato convenuto che l'avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai, ai fini dell'elezione da parte del Senato, sia pubblicato sul sito Internet istituzionale nella giornata di giovedì 21 marzo.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, nel giorno del trentesimo anniversario della morte di don Peppe Diana, è un onore per me ricordare in quest'Aula il suo esempio, che è diventato punto di riferimento per tutte le persone che hanno cara la cultura della legalità e la lotta alla mafia. Per amore del mio popolo non tacerò. Questo aveva detto don Peppino - come lo chiamavano tutti - tre anni prima di essere ucciso. Non lo fece mai, non tacque mai: con coraggio, per tutta la sua vita denunciò nomi, volti, numeri e pronunciò la parola «camorra» di fronte al mondo, smascherando quel castello di violenza e sottomissione che cementa i rapporti della criminalità organizzata. Scrittore intelligente, *scout* appassionato e vero alleato dei giovani, don Diana insegnava ogni giorno con la penna e con le azioni a ribellarsi alle catene imposte dalla mentalità mafiosa e a perseguire con tutte le forze, con tutta l'anima e con tutta la ragione, una vita libera, piena, giusta, nella legalità e nella trasparenza. A me non importa sapere chi è Dio, mi importa sapere da che parte sta. Così, non rinunciando alla provocazione, alla forza delle parole, dal pulpito come dagli editoriali a sua firma nel mensile «Lo spettro», invitava i confratelli e la Chiesa Chiesa tutta ad abbandonare la neutralità omertosa che spesso caratterizzava le istituzioni religiose e a denunciare le carenze dell'azione pastorale e sacerdotale e dello spirito di servizio alla comunità. Invocava nuovi modelli di comportamento, esempi concreti, omelie non reticenti, pratiche della solidarietà e dei valori etici e civili; essere, cioè - per usare di nuovo le sue parole non solo credenti ma credibili. Non risparmiava giustamente nemmeno le istituzioni civili campane, il cui parziale disfacimento aveva consentito l'infiltrazione camorristica a tutti i livelli, riempiendo un vuoto di potere dello Stato che nelle amministrazioni periferiche era caratterizzato da...

nella stessa parrocchia di Casal di Principe, aprendo le porte a chi troppo spesso se le era viste chiudere davanti: persone di origine africana prima e giovani donne dell'Est Europa in seguito, strappandole alla tratta della prostituzione. Aveva compreso che dove regnano povertà, emarginazione, disoccupazione e disagio, quindi anche quando si smantellano, indeboliscono o semplicemente non si attuano protocolli di accoglienza e inclusione delle persone migranti, è facile che le mafie si infiltrano. Stiamo seguendo la vicenda del liceo di Partinico a Palermo che non riesce a intitolare la scuola a Peppino Impastato per l'opposizione del Comune e per la contrarietà di una parte degli studenti: una questione che rischia di deteriorare i valori dell'antimafia, l'esempio di chi ha pagato con la vita per essersi opposto alla criminalità. Presidente, tra due giorni, il 21 marzo, sarà la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: una ragione in più per ricordare don Peppe Diana, perché i valori che trasmette la sua vita alle nostre comunità, a partire dal rifiuto dell'individualismo e delle ingiustizie, dalla lotta contro contro la camorra, sono gli anticorpi che servono al Paese per ribellarsi alla criminalità organizzata e per costruire una cultura della legalità e della responsabilità.